Senatori, è con profonda commozione che desidero esprimere a nome mio personale e di tutta l'Assemblea sentimenti di forte vicinanza e cordoglio ai familiari, ai colleghi e agli amici del dottor Giancarlo Salone, scomparso domenica scorsa a soli Giovane consigliere del Senato della Repubblica, il dottor Salone era diventato in poco tempo una delle principali figure di riferimento del Servizio delle Commissioni; questo non solo per le sue indiscusse competenze nelle materie giuridiche ed economiche, non solo per lo scrupolo, la professionalità e la dedizione quotidianamente dimostrati al servizio di questa istituzione, ma anche per la sua non comune capacità di ascoltare e di comprendere le esigenze di tutti, senatori, personale dei Gruppi, colleghi, cercando di trovare sempre una soluzione ai tanti problemi e alle tante questioni che caratterizzano ogni aspetto dell'attività parlamentare. Prezioso è stato, inoltre, il suo impegno come segretario e portavoce dell'Associazione consiglieri parlamentari in un periodo particolarmente delicato di riforme e di interventi che hanno interessato il personale del Senato. Studioso appassionato, persona mite e riservata, il dottor Giancarlo Salone era universalmente apprezzato anche per la sua spontanea umanità e un carattere estremamente gentile e dialogante. Fino all'ultimo abbiamo sperato e pregato che il dottor Salone potesse risvegliarsi dal coma e riprendersi dalle terribili conseguenze del tragico incidente stradale di cui era stato vittima un anno e mezzo fa. Con Giancarlo Salone ci lascia un consigliere di grande valore, un uomo perbene, un amico sincero e leale. In ricordo del dottor Giancarlo Salone, invito pertanto l'Assemblea a stringersi al dolore della mamma

*(M5S)*. Signor Presidente, sono rimasto favorevolmente stupito dalla proposta del senatore Candiani, tanto che dichiaro che il mio voto sarà favorevole cercherò di articolare un minimo la richiesta dal senatore Candiani.

aspettando anche le decisioni del Parlamento, in funzione di quelle che possono essere delle aperture o delle chiusure. Noto che anche i colleghi della Lega convengono e questa volta mi trovo favorevole non comprendo quale sia il motivo del brusio di fondo, quasi a contestazione. Stiamo affrontando un tema che è stato proposto da componenti dell'opposizione. Lasciamo che l'intervento del senatore

spiega) ci aveva proposto di esaminare le mozioni riguardanti gli spostamenti prima della riunione dei capi delegazione, proprio perché, con il voto del Parlamento, voleva condizionare

intervenire sull'ordine dei lavori. Faccio una richiesta ai colleghi della Lega, proprio per non evidenziare disinteresse e anche mancanza di coerenza rispetto alle posizioni prese durante la riunione della Conferenza dei Capigruppo di ieri, che ci ha trovato tutti concordi nell'identificare un calendario adeguato affinché la votazione sulle nostre mozioni e la conseguente presa d'atto da parte del Governo abbiano un senso compiuto. Chiedo ai colleghi della Lega di ritirare la proposta di inversione

che rendono ancora più strette le norme già previste dal precedente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre

Noi condividiamo la necessità di invitare tutti gli italiani a estrema prudenza. La prudenza deve essere esercitata in ogni circostanza. Purtroppo ci si può contagiare anche tra parenti o tra amici carissimi; il virus è estremamente egualitario e colpisce tutte le classi sociali, tutte le etnie, tutte le Regioni del nostro splendido Paese. Dunque non si può pensare, ed è molto pericoloso farlo, che tanto è Natale e allora non succede nulla. Pertanto, condividiamo facciamo nostro l'appello alla prudenza: si possono incontrare gli amici e i familiari ma non è indispensabile abbracciarsi, è opportuno stare comunque a una distanza decorosa e opportuna dalle persone. Già può essere una gioia rivedersi e trascorrere insieme qualche momento, in particolare per le persone isolate, per gli anziani o anche per i non anziani che vivono da soli, per i genitori separati e per i loro figli, che hanno rare occasioni di trascorrere insieme qualche momento. quello che non si può fare il 24 o il 25 dicembre lo può fare prima del 20 dicembre e dopo il 6 gennaio non ha senso. Intanto ci si può contagiare anche il 15 dicembre o il 10 gennaio,

Nelle altre circostanze, prima e dopo, è molto più difficile, in particolare per quanto riguarda le situazioni dei genitori separati lontani dai loro figli

per evitare situazioni di inutile discriminazione. Limitare al Comune gli spostamenti è una cosa scritta veramente da burocrati, anche poco informati. *(Applausi)*. Non c'è bisogno di essere tutti i giorni per le strade del nostro splendido Paese per sapere che ci sono

ma è estremamente inverosimile che gli affetti familiari (i genitori, i figli, i fratelli) siano residenti in quello stesso ristrettissimo La questione è cercare di limitare i contatti; verissimo, bisogna cercare di limitarli, ma non dimentichiamo che ci si contagia benissimo anche tra

di lunga portata (in molti casi, ma non sempre) implicano l'utilizzo di mezzi di trasporto pubblici (come treni, aerei e così via), dove ci potrebbe essere un assembramento. Ma, se si parla di spostamenti di pochi chilometri o di poche decine di chilometri, è evidente che andranno a piedi (in qualche caso bucolico e quasi ideale) oppure andranno con i mezzi propri, di conseguenza senza avere contatti con persone che non facciano parte della stessa famiglia. valutazione che avrebbe dovuto essere fatta da chi ha redatto e firmato il decreto-legge, cioè il Presidente del Consiglio e gli altri membri del Governo. Noi chiediamo di intervenire adesso; per la verità è già un po' tardi: sarebbe stato meglio farlo prima, perché le famiglie e le persone devono anche programmare i loro viaggi e devono cercare di far combaciare i loro momenti liberi. Arrivare al 15 dicembre è già tardi, ma meglio tardi che mai. Il decreto-legge è del 2 dicembre: se si fosse intervenuti quando il decreto-legge è stato

per evitare i tantissimi casi di quegli italiani che vivono a ridosso di confini di Provincia, consentendo degli spostamenti in quei giorni. Ricordiamo che certamente occorre adottare tutte le misure preventive rispetto al contagio, ma dobbiamo anche pensare in particolare alle situazioni

Il fatto di privare queste persone di questi momenti di gioia in un anno così difficile - pensiamo a quante famiglie sono state colpite da lutti, sia a causa del Covid che per altri motivi naturalmente non fa bene neppure alla salute. Non è una questione di buoni sentimenti: lo dicono eminenti immunologi,

volentieri, in modo da consentire alle persone in questi giorni molto particolari di un anno molto difficile di poter essere nuovamente vicine ai loro cari.

del nostro vivere civile. Parto da qui perché bisogna imparare ad andare oltre il *derby* tra aperturisti e rigoristi. Qui affrontiamo il tema della complessità: dentro un mondo sempre più integrato, si il Covid, una sfida che in qualche modo mette in discussione tutte le democrazie occidentali, possa essere affrontato tenendo conto proprio della sua complessità e nella sua interezza

conquiste storiche, magari date per scontate, mentre in questo momento tutti - soprattutto le nuove generazioni - comprendiamo quanto sia delicato andare ad incidere sul tema della mobilità tra le persone e sugli affetti più profondi. A maggior ragione, per le società liberali è tutto maledettamente più complicato: parliamo infatti di società articolate in diversi livelli di governo, società in cui bisogna convincere le opinioni pubbliche e in cui serve un processo di accompagnamento. Per questo è fondamentale che non ci sia solo il ruolo del Governo tecnico-scientifico ma debba esserci un protagonismo del Parlamento, perché noi siamo i rappresentanti di quell'opinione pubblica che ha bisogno di essere convinta, che deve comprendere le norme. Questo è uno dei passaggi fondamentali per le società liberali, rispetto ad altri sistemi di potere. Parto da qui, perché è evidente che abbiamo due strade davanti a noi. O ci rassegniamo agli automatismi del

anche conflittuale (ciò è però inevitabile, perché dentro le società liberali anche gli organismi tecnici risentono di una complessità di visioni e di opinioni diverse), oppure proviamo ad accompagnare il lavoro dell'Esecutivo con un necessario dibattito politico, esaltando il ruolo del Parlamento in termini di indirizzo politico rispetto alle scelte che devono essere prese. Quindi, o ci rassegniamo a mere decisioni tecniche o le proviamo a filtrare il ruolo politico e le prerogative di noi parlamentari. Questo è uno dei punti fondamentali: noi questo ruolo abbiamo deciso di esercitarlo, con le indicazioni che daremo rispetto alle scelte che dovrà fare il Governo in queste ore. Quindi, riconosciamo il ruolo, la difficoltà e la fatica del Governo, dentro una democrazia liberale come la nostra (una fatica simile a quella che stanno facendo altri Paesi europei), ma allo stesso tempo rivendichiamo il nostro ruolo di parlamentari che possono dare delle indicazioni.

il numero di positivi sui tamponi fatti si attesta intorno al 10 per cento, ma probabilmente ci saremmo aspettati un calo ancora più consistente. Quindi è giusto tenere alta la guardia, soprattutto perché entriamo in un periodo in cui potranno crescere le influenze stagionali, anche se i dispositivi quest'anno ci portano ad essere più protetti. È evidente che non possiamo abbassare la guardia, perché abbiamo da tenere in sicurezza e non mandare sotto *stress* le strutture sanitarie,

la lentezza con cui la curva scende ci impone grande attenzione, soprattutto nei giorni di festa. Dall'altro lato c'è il principio della progressività. Sento a volte un dibattito, anche estremamente facile ordine al fatto che negli altri Paesi agiscono diversamente. In realtà tutti i Paesi affrontano le stesse dinamiche, con le stesse difficoltà. Il dibattito in Germania è stato emblematico: in tre giorni hanno cambiato tre posizioni. Prima hanno detto che avrebbero fatto il *lockdown* dopo le festività natalizie, poi hanno detto che inizierà

la difficoltà delle democrazie occidentali nel costruire il consenso e nel convincere le persone e l'opinione pubblica a rinunciare alle libertà fondamentali, frutto della conquista delle generazioni precedenti. È infatti qualcosa che ha ha a che fare con il DNA stesso di un popolo, con la sua identità più profonda, e quindi noi giochiamo anche tenendo conto di questo aspetto. C'è poi il principio dell'equità e della ragionevolezza, un tema che come Partito Democratico abbiamo posto due settimane fa.

che le suddette misure siano vissute e percepite dai cittadini non solo come necessarie, ma anche come giuste e ragionevoli (presupposto indispensabile ai fini del loro pieno rispetto)».

quella fatica che - mi rendo conto - bisogna compiere per provare a tenere insieme tutti i principi, ivi compreso quello secondo il quale la norma come comprensibile e ragionevole da parte dell'opinione pubblica. Questo è un ulteriore sforzo, ed è il motivo per cui avevamo posto la necessità di evitare difformità di trattamento tra i piccoli e i grandi Comuni. Non voglio approfondire questo passaggio, che abbiamo davanti è tenere insieme tutti questi aspetti e principi. Quindi, prudenza, rigore, tenere alta la guardia rispetto all'evoluzione del quadro epidemiologico, progressività (quindi essere pronti ad adattare le misure a seconda del cambiamento del quadro epidemiologico),

che nel momento in cui si prendono misure fortemente restrittive ci sia anche la necessità di ristorare tutti quegli esercizi commerciali e tutte quelle persone che vengono penalizzati dalle stesse. Questo deve avvenire nello stesso momento, proprio per spiegare, raccontare, dare l'idea all'opinione pubblica che siamo consapevoli che, ogni volta che facciamo una scelta necessaria, fondamentale per la salute delle persone,

la necessità di mettere in campo misure restrittive: che il Governo possa farlo tenendo conto dell'andamento della curva epidemiologica e della necessità non solo di essere pronti, con il prossimo anno, a tenere sotto controllo ed evitare lo stress delle strutture sanitarie, ma di avere il sistema sanitario italiano preparato per il grande piano di vaccinazioni di massa nel nostro Paese. Governo a rivalutare le misure, con particolare riferimento agli spostamenti nelle giornate del 25 e del 26 dicembre, sulla base della più rigorosa analisi delle evidenze scientifiche fornite dal comitato tecnico-scientifico, e allo stesso tempo - come dicevo poc'anzi - nell'eventualità di nuove restrizioni, a prevedere misure di ristoro economico proporzionate alle perdite di fatturato anche nei confronti di quelle attività per le quali attualmente è prevista Il nostro ruolo è al fianco del Governo nel prendere le decisioni migliori, ma aiutandolo con il racconto di quanto ascoltiamo ogni giorno sui territori dalle imprese, dagli esercizi commerciali, dalle nostre famiglie.

non ci saranno gli abbracci calorosi, le riunioni di famiglia, che molto spesso erano momento di straordinario incontro con i cari trasferiti altrove. Non ci saranno neanche i tanti regali, le tavole imbandite, perché molti stanno vivendo un periodo di grave crisi economica. Ci apprestiamo a vivere il Natale dei nostri bisnonni, dei nostri nonni: un Natale essenziale, semplice, dove i piccoli gesti assumono un immenso valore. Peccato, però, che le limitazioni agli spostamenti in alcuni contesti urbani ostacolino la possibilità del ricongiungimento familiare durante le festività. A tal riguardo, mi chiedo semplicemente il motivo per il quale un cittadino romano abbia la possibilità di muoversi all'interno di un'area che si estende, come diceva anche il collega Malan, per 1.287 (percorrendo così anche 50 chilometri all'interno del proprio Comune), mentre un cittadino di un piccolo centro italiano sia costretto a spostamenti limitati, spesso separato dal resto della famiglia. Credo sia giusto discuterne oggi ed è necessario trovare una soluzione, un criterio proporzionato e oggettivo, al fine di consentire uguale possibilità di spostamento a tutti gli italiani. Faccio l'esempio dei nonni, magari rimasti soli dopo la dipartita del compagno o della compagna della vita, costretti a vivere in solitudine in questi mesi di chiusura, con poca interazione sociale, limitata magari ai soli momenti della spesa settimanale, anch'essa spesso resa impossibile per la mancanza in questi piccoli centri delle attività commerciali; è giusto, per via di una divisione sulla carta, che non potranno godere della presenza dei nipoti durante il giorno di Natale? Penso poi ai padri e alle madri separati, che non potranno raggiungere il figlio per consegnare il regalo il giorno di Natale.

la densità abitativa in questi luoghi non è altissima perché negli anni le famiglie si sono separate e spostate nelle zone urbane, lasciando zie e nonni nelle aree più periferiche che si sono tramutate in luoghi del cuore. Allo stesso tempo, però, è giusto pensare alla tutela della salute, al miglior metodo per prevenire i contagi. Non abbiamo i paraocchi, basta dare un rapido sguardo ai dati per comprendere che purtroppo i momenti difficili non sono terminati. Siamo uno dei Paesi che ha subito e sta subendo un attacco sanitario ed economico tra i più pesanti in Europa. Questa pandemia ci ha catapultato nell'anno più duro per numero di vittime dal 1944, quando ancora si vivevano i duri anni della Seconda guerra mondiale. Alla luce di ciò, la cautela è fondamentale; è di vitale importanza imparare dalla storia e dagli errori commessi. È però triste constatare che il Governo non abbia appreso nulla dall'ultimo tragico anno trascorso. Siamo arrivati impreparati alla seconda ondata, mentre pensavamo ai banchi a rotelle

ricorso alle strutture sanitarie pubbliche che, anche per i dodici anni di commissariamento, sapevamo avere un limite strutturale. È inaccettabile. Non si è lavorato per dotare le Regioni di sufficienti tamponi rapidi, così da mirare a *screening* veloci della popolazione e non si è pensato ancora di lavorare per individuare dei posti dove collocare i contagiati al fine di evitare la trasmissione del virus all'interno del nucleo familiare. Insomma, una vera disfatta. Era ottobre quando, annunciando le nuove misure, si dichiarava di doverlo fare per scongiurarle di nuovo durante le festività natalizie. stata scelta la strada della prevenzione e che volessero tutelare ancora la nostra economia (solo per i ristoranti chiusi è stimata una perdita di 720 milioni di euro nei giorni di festa); invece no, siamo ancora una volta qui a brancolare nel buio, a rincorrere il virus*,* accumulando sempre più ritardo. Temo che arriveremo impreparati anche sulla questione del piano vaccinale. Spero che presto queste mie parole vengano smentite da fatti concreti; significherebbe che la somministrazione del vaccino sarà partita senza intoppi e soprattutto senza commettere gli errori di qualche mese fa con il vaccino antinfluenzale. Bisogna però constatare che sono diverse settimane che il commissario Arcuri, delegato dal Governo alla gestione delle più delicate questioni legate all'emergenza in corso (neanche fosse dotato di superpoteri), discute in merito alla somministrazione dei vaccini. Esprimo le mie preoccupazioni in merito alle tempistiche con cui questa situazione si risolverà,

oggettivi, uniformi e chiari per gli spostamenti il giorno di Natale, nonché aiuti concreti, rapidi e commisurati a chi sta soffrendo anche economicamente. Il secondo appello è alle famiglie, affinché siano consapevoli del grande rischio cui si va incontro.

tutte le proposte del nostro Gruppo sono entrate - e di questo siamo contenti - nella mozione unitaria di maggioranza, cui chiedo anche ufficialmente di aggiungere la mia firma. Avevamo chiesto già nei giorni scorsi tre punti essenziali: coerenza, dati scientifici certi, programmazione. Il *caos* generato nei giorni scorsi, la confusione e anche - mi dispiace dirlo un comitato tecnico-scientifico che si era diviso e spaccato anche sulla certezza dei dati epidemiologici aveva mandato davvero in confusione i cittadini e le famiglie e non solo coloro

i ristoratori, i commercianti, coloro che ovviamente necessitano di avere una programmazione chiara anche rispetto ad alcune indicazioni che erano state già date (penso al pranzo di Natale, e al pranzo di Capodanno in modo particolare).

e non su spaccature anche del mondo scientifico e chiaramente massima tutela della salute dei nostri cittadini, perché è chiaro che questo è un punto fondamentale. Siamo preoccupati, come tutti, dei dati di questi giorni e anche delle immagini che abbiamo visto sui telegiornali, delle foto che sono apparse su molti giornali, ma non possiamo vivere ogni giorno con un'incertezza, soprattutto quando questa poi si manifesta anche all'interno del Governo e del Parlamento. È per questo che sin dall'inizio abbiamo chiesto di avere una visione chiara,

rafforzare le nostre strutture ospedaliere, sostenere e aiutare un personale sanitario infermieristico e tutti gli operatori sociosanitari che hanno bisogno di essere supportati, perché fanno turni massacranti e sappiamo che molte strutture sono al collasso. Abbiamo anche detto in maniera chiara - lo ha

hanno bisogno di lavorare e di riprendere in mano questo Paese anche dal punto di vista economico. Chiudo con un accenno ai ristori. Anche a tale proposito è stato scritto in maniera chiara - e lo abbiamo detto più volte come Italia Viva è evidente che se si dovesse andare verso una linea più rigorosa, con più misure restrittive, dovremmo prevedere immediatamente ristori adeguati alla perdita di fatturato anche di coloro che in questi giorni, come ristoratori, avevano già fatto acquisti per preparare

Chi l'avrebbe mai detto? Una cosa impensabile un anno fa. Inutile nascondersi che in quest'ultimo anno la nostra vita è stata stravolta. Ci siamo scoperti fragili e siamo stati chiamati a dover valutare l'importanza di una scelta rispetto ad un'altra con l'unico scopo di tutelare la vita di tutti. Abbiamo perso quasi 66.000 nonni, genitori, figli, zii, cugini, amici. Ogni cosa, ogni parola, ogni decisione che prendiamo oggi e che abbiamo preso negli ultimi mesi ha avuto questo macigno sulle nostre menti. Tra quelle persone che non ci sono più c'erano anche 259 medici, infermieri e operatori sanitari che hanno scelto di mettere la cura degli altri davanti alla propria. Noi siamo parlamentari e abbiamo il dovere di rappresentare - in questo caso anche difendere - la salute e la vita dei nostri concittadini. L'istanza di protezione è già assolta dai provvedimenti governativi, sempre precisi, puntuali e commisurati rispetto alla situazione del Paese. Quindi attenzione, colleghi, perché pur plaudendo alla posizione del Presidente del Consiglio Conte, che ha sempre voluto salvaguardare la prerogativa del Parlamento di poter indirizzare l'azione governativa, sento il dovere di sottolineare l'importanza di valutare bene ogni nostra iniziativa o votazione. Infatti ogni scelta deve essere supportata da elementi concreti, e soprattutto, da una base scientifica solida per evitare decisioni che poi si possono ripercuotere come un *boomerang* sulla stessa pelle degli italiani. È chiaro che ogni decisione presa dal Governo fino ad oggi sia stata assunta solo dopo aver consultato approfonditamente il comitato tecnico-scientifico, gli attori sociali e le Regioni. La nostra azione parlamentare deve essere immune, per quanto difficile, da istanze personalistiche o provenienti da un collegio elettorale o da altro che inevitabilmente può condizionare il giudizio. Non si può prescindere dal quadro epidemiologico attuale e dalla sua evoluzione quotidiana e futura. Per questo sono convinto sia importante innanzitutto tornare a strutturare il nostro giudizio e il nostro lavoro attorno al criterio fondante della responsabilità, una parola ripetuta più volte in questi mesi di pandemia. A volte ne abbiamo anche abusato perché credo che la maggioranza dei cittadini sia stata encomiabile nel rispettare i dettami precauzionali nella lotta contro il virus. Proprio per questo credo anche che non si debba stigmatizzare eccessivamente chi, ad esempio, seguendo comunque le regole ha inteso visitare i negozi dei centri cittadini negli ultimi giorni. Dall'altro lato, però, credo anche che lo stracciarsi le vesti di fronte l'ultimo DPCM che ha voluto evitare grandi rischi, bloccando gli spostamenti a Natale, a Santo Stefano e a Capodanno, sia estremamente eccessivo. Nelle mozioni odierne (e sono contento che si sia trovato un accordo di maggioranza) si vuole affrontare un problema relativo ai piccoli Comuni che sembrano penalizzati rispetto ai gradi. Qual è la soglia oltre la quale impedire gli spostamenti tra Comuni? una decisione molto difficile da prendere e, credetemi, ci sarà sempre qualcuno che vorrebbe alzare l'asticella. Tre giorni: il Governo ha chiesto praticamente solo tre giorni di sacrificio più accentuato nelle due settimane di festività. Tra l'altro, ha anche previsto che gli spostamenti per necessità, lavoro o motivi di salute, siano in ogni caso salvaguardati. Colleghi, smettiamola quindi di raccogliere esempi casuali, estremizzati e del tutto strumentali. Se ci sono persone anziane che abitano da sole e non sono autosufficienti, saranno accudite. Si tratta ovviamente di una casistica già inserita all'interno delle situazioni di necessità, e non c'è bisogno di strumentalizzare le persone in difficoltà. Certo che se all'interno dello spostamento tra Comuni piccoli si intende liberalizzare pranzi, cene e baldoria, allora il problema non è il Governo né il virus in sé. Le festività legate al periodo natalizio fanno parte della nostra tradizione Ognuno di noi ha ricordi indelebili della propria infanzia, quando ci bastava veramente poco per sentire il calore degli affetti. Provengo da una famiglia numerosa, siamo nove fratelli, molto legati ad altrettanti numerosi cugini, e quando ci si riuniva per le festività erano veramente momenti di gioia pura e genuina. Ora siamo cresciuti e i nipoti sono già venti. Immaginate i nostri Natali quanto sono stati trafficati tra tombole, calze, chiacchiere al tepore del camino. ottantacinque anni ed è ancora piena di energie *(Applausi);* ha compreso che quest'anno non potremo farle visita e, proprio per poter rivivere in un prossimo futuro questi momenti di calore familiare, dobbiamo tutti fare questo sacrificio. Ha compreso, non si è data per vinta e ha preparato per tutti tortellini e torte, conservati nel congelatore per quando potremo raggiungerla in sicurezza. È in grado di utilizzare la videochiamata e la introdurremo via Zoom a una tombolata a distanza: anche questo è un modo per non lasciarla sola. Colleghi, a molti queste norme prudenziali possono apparire un limite insopportabile, ma non c'è nulla che possa essere messo davanti al rischio di nuocere agli altri, ai nostri genitori, ai nostri nonni. Personalmente, trovo che quest'anno anche il giorno di Natale potrà lasciarci dei momenti preziosi. Magari, pensare intensamente a chi non è temporaneamente con noi ci farà apprezzare maggiormente il tempo che poi passeremo di nuovo insieme. Credo che il pensiero più profondo del Natale possa essere veramente quello di amare i nostri cari. Se normalmente lo facciamo con calore e in compagnia, questa è la volta di dimostrarlo con una faticosa, ma doverosa rinuncia. La cosa più importante è che ogni scelta avvenga su base scientifica, sulla base dei dati, non su onde emozionali; altrimenti, dovendo seguire quelle, sono sicuro che tutti noi vorremmo sentire per la casa le urla dei nostri nipoti, dei nostri figli, sederci a tavola, abbracciarci, condividere così il Natale come abbiamo sempre fatto. Manca un ultimo sforzo e non possiamo vanificare quanto fatto finora; non possiamo mettere a rischio chi più amiamo.

Signor Presidente, penso che un fondamento obiettivo del rispetto delle norme sia l'obiettiva ragionevolezza e soprattutto che le persone possano condividerle ed anche comprenderle. Penso che una normativa, almeno come è stata prevista fino ad oggi, che anche per il ricongiungimento degli affetti - e non solo per quello, ma anche per gli spostamenti - nei giorni di festività più importanti

quindi ci debba essere un criterio di omogeneità sul territorio, perché se c'è un pericolo di contagio, di assembramento, nelle famiglie o nei ristoranti, dove

L'Italia è soprattutto un territorio di piccoli e medi Comuni, una periferia e una provincia che spesso si sentono bistrattati e dimenticati, anche a torto (ma alcune volte a ragione).

omogeneità sull'intero territorio nazionale. Naturalmente, la cosa deve essere comprensibile alle persone perché la norma per essere rispettata deve essere comprensibile. Noi abbiamo anche il dovere di fare scelte dolorose, difficili e necessarie, soprattutto a tutela della salute delle persone. La tutela della salute delle persone è omogenea sul territorio nazionale e, quindi, i criteri che devono guidare

al turismo, all'accoglienza, alla ristorazione e alle piccole e medie imprese che avranno a soffrire in misura maggiore rispetto a questa situazione. È chiara la

perché le situazioni che possono essere prodromiche al propagarsi dell'influenza o del virus del COVID siano molto contenute. Però chi abita nei piccoli e medi Comuni della nostra Italia

intervengo oggi non solo in qualità di senatore, ma soprattutto in qualità di sindaco di un Comune con poco più di 10.000 abitanti. Come forse qualcuno di voi sa, ho l'onore di vestire la fascia tricolore del Comune di Orzinuovi in provincia di Brescia. Il Comune è stato duramente colpito durante la prima ondata di pandemia dello scorso marzo, che ci ha costretto a registrare più di 120 decessi su 12.000 abitanti.

Tuttavia, da sindaco, non posso che esprimere la mia preoccupazione in merito alle prossime restrizioni previste per le festività natalizie. Sia ben chiaro che la priorità per tutti noi è la salute e, considerando ciò che ho vissuto come primo cittadino

Ciò nonostante sono convinto, come tutti gli altri sindaci che potrei oggi rappresentare, che tutelare i più deboli significa permettere loro di poter passare un Natale a fianco dei propri cari, nel massimo rispetto di ogni indicazione contro il Covid. Durante quei giorni so per certo, colleghi, che molte persone non potranno contare sulle assistenze domiciliari a cui solitamente fanno affidamento. Sappiamo bene tutti che non è la medesima cosa vivere in una città capoluogo di Provincia o in un grande centro abitato rispetto invece a vivere in un piccolo Comune. A questo poi va aggiunto che molte persone, spesso anziane, vivono sole con i figli lontani molti chilometri. Si pensi pertanto a una serie di provvedimenti che possano tutelare la salute dei più fragili sotto ogni punto di vista; si pensi a soluzioni che possano garantire sicurezza della salute, ma anche la salute emotiva e sociale. Riteniamo che sia nostro compito e dovere farlo.

prima di entrare nel merito del decreto di Natale vorrei fare un piccolo passo indietro, a quando lo scorso marzo il Covid ha stravolto le nostre vite. Ovviamente in un primo momento ci siamo trovati tutti spiazzati da questa situazione nuova e indecifrabile e ciò ha portato il Governo a prendere decisioni emergenziali sull'onda della fretta e della paura e noi, le opposizioni, a tollerare scelte che già con il senno di allora, ma certamente con il senno di poi, si sono rilevate spesso azzardate e incongruenti. Gli italiani hanno dovuto affrontare una situazione con limitazioni frustranti per il nostro modo di fare e di essere. Persino la Pasqua, momento tradizionalmente di resurrezione e luce è purtroppo stata buia e dolorosa. Ora si prospetta un avvicinamento al Natale, il cui travaglio e parto rischiano di essere - ahimè - altrettanto dolorosi e bui. Dopo ormai dieci mesi di pandemia non è più possibile affrontare la situazione proponendo soluzioni di dubbia utilità, mentre basterebbe solo un po' di sano e vecchio buon senso. Per questo anticipo che presenteremo un testo 2 della mozione, dove, oltre alla richiesta di un maggior buon senso per quanto riguarda gli spostamenti, chiederemo anche un risarcimento - e sottolineo risarcimento e non ristoro per la perdita del fatturato del 75 per cento qualora alcune attività commerciali dovessero subire danno dalle scelte del Governo. Inutile spargere sale, infatti, sulla ferita dei miliardi spesi per i banchi a rotelle o sui fallimenti dei vari *bonus*: un'apoteosi di spese senza senso uno spreco assurdo, così come non ha alcun senso incentivare le spese con il *cashback* e la lotteria degli scontrini e poi meravigliarsi che gli italiani facciano quello che è stato chiesto loro, ovvero spendere soldi nei negozi fisici per far ripartire l'economia. A proposito di buon senso, ne basterebbe veramente poco per capire che c'è un'evidente contraddizione nel permettere a milioni di cittadini romani di percorrere chilometri e chilometri, all'interno quindi del loro vasto Comune, e costringere le poche anime del Comune di Abetone Cutigliano nella montagna della mia Pistoia, oppure di Volturara Appula, che conta 392 abitanti, a restare nel loro piccolo recinto. Vedete, colleghi, non è solo una questione di fare scelte approssimative, ma di arrecare danni lapalissiani ai nostri concittadini. Basti pensare che spesso in queste piccole realtà che ho citato mancano addirittura le attività commerciali. Non si può nemmeno fare un piccolo dono di Natale, a meno che un pacco di farina non si voglia considerare un dono di Natale. Insomma, io non so come vengano fatte le

torto a nessuno), io ritengo che questa, come moltissime altre iniziative prese dall'inizio di questa emergenza, sia il risultato di un completo allontanamento della politica dai cittadini e dalla loro vita reale. Mi sembra che non abbiate contezza del tessuto sociale su cui calano come scure i vostri provvedimenti presi notte tempo; che non conosciate la struttura morfologica ed orografica del nostro Paese, ricco di Comuni e frazioni con meno di mille abitanti. Sembra, e forse è davvero così, che non sappiate che ci sono genitori separati, cittadini fuori sede, non solo per studio ma anche per lavoro, costretti a stare lontani dalle proprie famiglie per tutto l'anno e che aspettano il giorno di Natale per stare insieme. La convivialità, lo stare in famiglia, le tradizioni non sono vizi o vezzi ai quali i cittadini non vogliono rinunciare per capriccio, ma sono parte integrante della nostra identità. Colleghi del Governo, io credo fortemente alla prevenzione e alle precauzioni. Condividiamo, come ha detto il senatore Malan, la prudenza. Per cercare di facilitare e velocizzare la ripresa di tutti, oltre che la prudenza, anche sapere cosa si sceglie per i propri cittadini. Quando abbiamo chiesto loro dei sacrifici, i nostri cittadini sono stati bravi. Non è vero che non hanno rispettato le regole. Gli italiani sanno rispettare le regole; paradossalmente, è vero il contrario: le sanno rispettare anche troppo, ma hanno necessità di avere regole certe, non schizofreniche, e che il perimetro di queste regole sia definito dal buon senso. Invece, l'approssimazione e la superficialità di molte, se non di tutte, le iniziative prese da questo Governo non hanno fatto altro che aumentare la loro confusione. Anche in questo caso, sarebbe bastata, forse, la diligenza del buon padre o madre di famiglia. Questa può venirvi in aiuto per cercare di proteggere in tutti i modi i nostri concittadini, senza snaturare le più elementari libertà. Certo, per fare questo si deve conoscere il proprio popolo; sapere quali sono le esigenze che lo caratterizzano e prendere, in base a questo, le decisioni migliori. a mio avviso, è il più grave errore di questo Governo: non avere dimostrato la dovuta sensibilità verso le priorità degli italiani. Ascoltateli e diamo loro un buon Natale.

dette dall'*ex* procuratore Nordio. Tutti i provvedimenti, anche quelli più radicali, possono essere giustificati in una situazione di emergenza, a patto, però, che siano razionali. Molte misure prese dal Governo per contrastare la pandemia appaiono irrazionali. Ad esempio, partiamo dal fatto che sembra che i ristoranti siano in sicurezza a mezzogiorno ma non lo siano, invece, la sera per la cena. Questo non lo capiamo. Si chiudono i centri commerciali nei weekend e poi ci si stupisce che gli assembramenti avvengano tutti davanti al piccoli negozi nei centri delle città. Si parte in pompa magna col *cashback*, invitando i cittadini ad andare a spendere. Spendete: 10 transazioni entro la fine del mese (siete partiti l'8 dicembre) e vi possiamo ridare indietro il 10 per cento. Quindi, un invito ad andare nei negozi e poi si colpevolizzano i cittadini perché ci sono andati. Anche qui, non capiamo la ragionevolezza di certe norme. Si dà il *bonus* vacanza, ma poi, alla fine, in vacanza sostanzialmente non ci si può andare ed è vietato. A Natale, a Santo Stefano, a Capodanno sono vietati gli spostamenti. Nelle grandi città, però, ci si può spostare senza problemi, con un raggio chilometrico molto elevato, se pensiamo alle metropoli come Roma, Milano, Napoli, Torino e le città metropolitane.

Che trovata! Così, tutti assembrati sui pochi treni e aerei che ci sono. Complimenti!

a un sindaco della Brianza: «Buongiorno sindaco, sono una cittadina residente a Lazzate, ma domiciliata a Lentate sul Seveso. Mi permetto di scriverle per raccontarle cosa è capitato alla mia famiglia in questo 2020, un anno da dimenticare. Noi siamo residenti a Lazzate da qualche anno; abbiamo comprato una casa in cui abbiamo vissuto io, mia madre, mio padre e mia sorella. Purtroppo il 2 gennaio un infarto ha colpito mio padre, che ci ha lasciato, e il 9 luglio un tumore fulminante ha portato via anche mia madre.

Io ho un fidanzato con cui vivo a Lentate e mia sorella vive sola a Lazzate con i nostri cani. Ieri sera» - la lettera si riferisce al giorno dopo l'emissione del DPCM «ho sentito il nuovo DPCM e, come mi aspettavo, mi è crollato il mondo addosso. In un anno terribile come questo, come posso pensare di poter passare il Natale senza quello che resta della mia famiglia? Chi governa non sa cosa succede nelle famiglie, non sa cosa voglia dire passare una festività con due lutti sulle spalle e in completa solitudine. Sono veramente a terra». Lei, sua sorella e il fidanzato: tre persone che non si possono vedere perché abitano in due Comuni che sono limitrofi. Però a Roma, a Milano e in altre realtà ci si può vedere anche in dieci, perché chiunque si può spostare. Dov'è, dov'è, dov'è,

le festività del Natale, a cui siamo molto legati, sono un momento importante di condivisione, in cui famiglie e amici si ritrovano per trascorrere del tempo insieme. Purtroppo quest'anno non potrà essere così, è inutile girarci intorno. Sappiamo benissimo che non stiamo vivendo tempi normali; siamo in piena pandemia. Una crisi sanitaria ci ha fatto perdere oltre 65.000 concittadini: nonni, genitori, figli, colleghi di lavoro e amici. Ognuno di noi in questi lunghi undici mesi ha perso qualcuno di caro. Altri sono stati male e hanno vissuto giorni di terrore, con conseguenze gravi per la loro salute. Abbiamo avuto quasi 2 milioni di casi. Siamo in guerra, lo diciamo tutti da mesi. Adesso cosa vogliamo fare? Raccontarci che non siamo più in guerra perché è il giorno di Natale? Non possiamo commettere errori: è il patrimonio umano a subire un duro, un durissimo attacco a livello globale. È vero, negli ultimi giorni i provvedimenti si sono inaspriti; è successo in Germania, in Gran Bretagna, in Olanda, nello stato della California, nella città di New York, dove si è deciso di attivare il *lockdown* più rigido, a pochi giorni dal Natale, infliggendo un duro colpo per i commercianti e per i cittadini. Perché? Basta controllare la curva di crescita, per esempio negli Stati Uniti *post* Thanksgiving, una festività per loro importante, dove tutti si sono spostati da una città all'altra e da uno da uno stato all'altro per raggiungere i propri cari. Questi dati ci mostrano la pericolosità di aprire agli spostamenti di massa durante le festività di Natale. Le scelte sono politiche, è vero, ma sono scelte che devono avvenire su base scientifica. Capisco che la Lega, con il suo *leader* Salvini, che si rifiutava di indossare la mascherina qui in Senato (tra l'altro durante un convegno di negazionisti), potrebbe sottostimare tutto questo. Ma per esempio l'onorevole Gelmini, non più tardi di lunedì scorso, tuonava contro la folla per le strade, dicendo che dobbiamo assolutamente scongiurare una terza ondata di Covid in Italia, perché non la reggerebbe il nostro sistema sanitario e ancor meno il nostro tessuto economico, già duramente colpito dalla crisi. Così tuonava.

tutti i volontari che si stanno occupando senza sosta dei nostri malati Covid. Abbiamo sentito dire che i nostri anziani sarebbero restati soli, quando non è vero, perché già ora è previsto di potersi muovere per dare aiuto a una persona che ne ha bisogno. Questo di certo - sia ben chiaro - è lontano dalle tavolate natalizie cui siamo abituati, alle meravigliose famiglie riunite attorno allo stesso tavolo: ci sono famiglie due, tre o quattro nuclei familiari si riuniscono solo per le feste. Quest'anno purtroppo è pericoloso. È una sofferenza, lo è per tutti, ma non abbiamo altra scelta. In Italia questa pandemia è stata sin da subito gestita con tempestività. Il Governo ha potenziato la sanità; abbiamo messo in campo più di 12 miliardi, invertendo totalmente la drammatica tendenza dei tagli (ben 37 miliardi negli ultimi dieci anni). Contemporaneamente abbiamo sostenuto le imprese e i lavoratori in difficoltà: con il decreto ristori, votato proprio ieri in Senato, l'ultimo di una lunga serie, abbiamo stanziato 19 miliardi. Il presidente Conte ha fatto appello alla responsabilità di tutti gli italiani, invitandoli a tenere alto il livello di guardia, per non rischiare di rendere vani tutti gli sforzi e i sacrifici fatti fino ad ora e ritrovarci di nuovo con un'ondata di Covid-19 dopo le feste. In questi giorni abbiamo visto scene di assembramenti nelle città italiane, con le vie dei centri storici, dello *shopping* e dello svago che sono state invase. I cittadini, comprensibilmente stanchi dopo undici mesi difficili dall'inizio della pandemia, forse hanno ceduto, sperando in un ritorno alla normalità, mentre ogni nostro spostamento non necessario rischia ora di essere

poiché la loro salute va tutelata sempre, anche il giorno di Natale. Non dobbiamo cedere al desiderio di passare le feste con i nostri cari, se questo rappresenta per loro un rischio; abbiamo il dovere di tutelare i nostri genitori, i nostri nonni, i nostri fragili. Arriverà il momento degli abbracci, dei baci e dei festeggiamenti seduti intorno a grandi tavolate con parenti e amici, ma questo tempo non è ora. Sacrifichiamo questo Natale perché il sacrificio di ogni famiglia permetterà di poterne festeggiare molti altri tutti insieme. *(Applausi)*.

gli italiani hanno dato grande prova di sé nei mesi scorsi. Se siamo riusciti a ridurre il numero dei contagiati e dei morti, nonostante le difficili condizioni, lo dobbiamo in gran parte anche ai tanti di loro che, per mesi, si sono attenuti diligentemente alle regole più severe fissate dal Governo. Per questo credo che dovremmo dire grazie agli italiani per ciò che sono riusciti a fare, piuttosto che sgridarli in continuazione a causa dei pochi che non rispettano le regole. Gli italiani hanno alle spalle mesi di lutti, di sofferenze, in cui tutti hanno fatto tanti sacrifici. Tanti, troppi hanno conosciuto da vicino il Covid perché hanno perso persone care o perché si sono ammalati loro stessi in prima persona o, ancora, perché stanno subendo le cause economiche della pandemia. Non c'è persona nel nostro Paese che non viva uno stato di profonda ansia, per gli effetti provocati da questo maledetto virus. In una situazione così estrema e drammatica, il ruolo delle istituzioni diventa ancora più importante del solito, del solito, per mettere in campo misure volte alla tutela dei propri cittadini, ma anche per coglierne lo stato d'animo ed essere punto di riferimento, in grado di ispirare fiducia e rassicurare rispetto al futuro. Gli italiani, la nostra gente, sono già abbastanza provati non hanno bisogno di decisioni estemporanee, né tantomeno di scelte che cambiano in continuazione. Invece, purtroppo, è proprio ciò a cui stanno assistendo i nostri concittadini: famiglie, commercianti, lavoratori, persone che ogni giorno guardano il telegiornale e non sanno ancora se possono programmare qualcosa, da qui a dieci giorni. Ciò vale per il singolo, che magari ha già comprato il biglietto del treno, per trascorrere i giorni di festa con i propri genitori anziani, e vale anche per migliaia di imprese, che non sanno ancora se potranno offrire o meno la propria attività lavorativa; se potranno occupare o no i propri dipendenti; se devono rifornirsi dei prodotti necessari per lavorare o se invece rischiano di sprecare risorse preziose, per poi doverle buttare, perché si è sempre in bilico, con il dubbio che, da un momento all'altro, cambino di nuovo le regole. Proviamo a metterci nei panni di chi ha un'attività in proprio, un ristoratore o il proprietario di un bar: come devono regolarsi per i prossimi giorni di Natale, che spesso contribuiscono fino al 40 o 50 per cento del fatturato dell'intero anno? Non sanno come devono comportarsi e questa purtroppo è la verità. A neanche dieci giorni di distanza dal Natale, non li abbiamo ancora messi nelle condizioni di potersi organizzare. Come Italia Viva lo diciamo da tempo: siamo per riaprire, in sicurezza, con il rispetto delle precauzioni e delle regole di sanificazione via via prescritte; con l'aumento delle corse dei mezzi pubblici, adottando tutte le misure necessarie per evitare assembramenti. Se però la maggioranza dovesse preferire adottare delle misure più restrittive, ne prenderemo atto, ma lo si faccia affidandosi a dati certi, scientificamente provati, in modo coerente e dando indicazioni precise, senza decisioni contraddittorie o dovute alle immagini trasmesse dalla televisione. Anche perché, signor Presidente, cosa avremmo dovuto aspettarci dalle piazze e dalle vie dello *shopping* italiano, se non la vita che torna a riempirle, appena si rallentano le restrizioni? È normale, è umano e, soprattutto, è stato alimentato dalle stesse decisioni assunte dal Governo, nella misura in cui si è ripetuto per settimane chiudere in autunno per salvare il Natale. Si è detto per settimane che il Natale era da salvare e, per farlo, si è conseguentemente adottata una serie di limitazioni, più o meno stringenti, su base regionale, in base agli indici RT, cioè a quel parametro che indica la capacità dell'epidemia di espandersi. Si tratta di misure che hanno portato evidenti miglioramenti rispetto al numero dei contagi, tanto che l'indice di contagiosità RT, su base nazionale, a differenza di quello di altri Paesi, è sceso sotto la soglia critica di 1. Adesso non ci si può stupire se le persone, con le dovute attenzioni - la mascherina e la giusta distanza - scendono a passeggiare e vanno nei negozi. Abbiamo detto che vogliamo chiudere i centri commerciali, che vogliamo salvare i centri storici; abbiamo invitato la gente a recarsi di persona nei negozi, dicendo loro che, se comprano lì e non su Internet, avranno indietro una sorta di premio, il cosiddetto *cashback*, e adesso ci stupiamo se vanno in centro a fare acquisti, ossia se fanno ciò che noi stessi abbiamo suggerito loro di fare. *(Applausi)*. Ciò rischia di trasformarsi in una colossale presa in giro. È un atteggiamento che, come Italia Viva, non ci appartiene. Non siamo per la colpevolizzazione di quegli italiani che sono perfettamente in linea con le leggi che sono state loro prospettate, né siamo per assumere decisioni solo perché altri Paesi le stanno adottando. È vero che Germania, Olanda e Gran Bretagna, dopo mesi di scarse restrizioni, hanno predisposto nuove serrate alle attività economiche e agli spostamenti. Ma è altrettanto vero che tali decisioni sono state dettate da un contesto molto diverso dal nostro, in cui si è riscontrato un repentino aumento delle rispettive curve dei contagi e un peggioramento della pressione sulle loro strutture ospedaliere, da noi si è riusciti a scongiurare, grazie alle misure differenziate, adottate nelle settimane scorse nelle diverse Regioni. Ecco che adesso siamo a chiedere maggiore coerenza rispetto alle politiche che si intendono adottare. A nostro parere vanno evitati gli allarmismi, così come vanno evitati i repentini cambi di regole. Solo pochi giorni fa si era ventilata l'ipotesi di rimodulare l'ultimo decreto attraverso un allentamento dei vincoli sugli spostamenti tra Comuni sotto Natale, salvo poi profilarsi l'ipotesi opposta di un *lockdown* ancora più severo: tutte dichiarazioni che creano sconcerto tra la gente e danni all'economia. Ci fa piacere che la maggioranza tutta abbia convenuto di convergere sulla nostra proposta affinché le scelte del Governo in tema di chiusure vengano prese sulla base di dati scientifici oggettivi e trasparenti, garantendo ristori immediati a chi deve chiudere. Bisogna fornire elementi certi, in via preventiva, ai cittadini, ai lavoratori e alle imprese così che si possano organizzare per tempo. Bisogna dare tranquillità a tutti gli operatori economici dai quali si pretende la chiusura nella misura in cui gli si danno garanzie rispetto all'assegnazione di risorse adeguate a compensare le mancate entrate. Penso al mondo della cultura, alla ristorazione, al turismo, alle strutture alberghiere, ma anche a tutti quei liberi professionisti e a quegli esercizi e fornitori di servizi che non potranno lavorare. Lì sì che dovremmo prendere a modello Paesi come la Germania, dove il Ministro delle finanze ha annunciato che le attività colpite da serrata potranno chiedere fino a mezzo milione di euro di contributi a ristoro, appunto, dei mancati introiti: cifre che suonano inimmaginabili a pensarle come ristoro, ma che possono effettivamente corrispondere alle mancate entrate di aziende ben funzionanti. Signor Presidente, il Natale è di solito sinonimo di abbondanza: abbondanza di affetti, abbondanza di compagnia, anche abbondanza economica. Quest'anno, invece, il Covid ci costringerà, per forza di cose, a un Natale segnato dalla scarsità e dalla mancanza: mancanza dei propri cari, mancanza di vicinanza, mancanza di sicurezze per il futuro. futuro. È ancora più urgente, allora, che come Governo, come legislatori e come istituzioni cerchiamo di colmare il senso di spaesamento e di vuoto, assumendo per tempo scelte oculate e coerenti per garantire in tempi difficili il miglior Natale possibile per tutti. *(Applausi)*.

I cittadini non si misurano solo col virus e con le sue conseguenze economiche, ma anche con nuove abitudini che sono il frutto delle regole emanate ora dal Governo, ora dalle Regioni e dalle Province autonome, ora dalle ordinanze dei sindaci. Nessuno mette in discussione la loro importanza e il fatto che talvolta devono reagire in tempi brevi all'evolversi del quadro epidemiologico; ma perché siano accettate dalla popolazione, queste regole devono essere comprensibili e giuste, nel senso che i sacrifici devono essere distribuiti in maniera equa tra tutti i cittadini, e non devono cambiare continuamente. L'ultimo DPCM ha dato regole precise con riferimento anche al periodo natalizio: le persone si sono arrangiate con queste regole. In Sudtirolo - per esempio - abbiamo fatto un test di massa, al quale ha partecipato quasi il 70 per cento della popolazione, a cui è stato promesso che, se avesse partecipato in massa, saremmo diventati presto zona gialla. Ebbene, anche se abbiamo già da tempo i presupposti, diventeremo zona gialla domenica, e lunedì scatteranno le restrizioni del periodo natalizio. Le regole già restrittive non possono essere cambiate pochi giorni prima della loro entrata in vigore solo perché hanno spaventato le immagini dello *shopping* lo scorso fine settimana; non possono ulteriormente limitare persone che sempre si sono attenute alle regole solo perché alcune le hanno trasgredite. Dovete controllare di più e non inasprire le regole. Mi domando, infatti: cosa è cambiato da quando avete emanato il DPCM con le regole sul Natale? Niente, anzi, come previsto, tutta Italia è diventata zona gialla. Non c'è alcun motivo, allora, per cambiare di nuovo le regole. L'approccio di continui cambiamenti viene percepito come ingiusto, come viene mal tollerato anche il divieto di spostamento tra i Comuni intorno a Natale e a Capodanno. A Milano, Napoli o Roma vivono milioni di persone che possono incontrarsi e girare liberamente, ma in Italia ci sono anche 5.500 Comuni che hanno meno di 5.000 abitanti, di cui quasi 2.000 con meno di 1.000. Nei giorni attorno al Natale per chi vive in una grande città il divieto di spostamento non comprometterà minimamente la possibilità di avere interazioni sociali e di svolgere tutta una serie di attività; invece, genitori e nonni che vivono in un piccolo Comune non potranno neppure vedere figli e nipoti. Ma non è solo questo. Chi vive nel piccoli centri non potrà neppure fare una passeggiata in montagna all'aria aperta, quando invece chi vive a Roma potrà comunque spostarsi su un territorio grande più di 1.000 chilometri quadrati. Penso che ci siano situazioni molto più pericolose di una passeggiata all'aperto nella diffusione del virus: nutrendosi dell'interazione e della vicinanza tra le persone, sono i centri a maggior densità quelli che dovrebbero destare preoccupazione e non i luoghi dove c'è una casa ogni 500 metri, anche se parliamo di due Comuni diversi. Non a caso, in nessun altro Paese europeo si prevede il divieto di uscita dal proprio Comune durante il periodo natalizio. Tante misure adottate finora negli altri Paesi europei sono uguali a quelle italiane, dalla chiusura di bar e ristoranti, al coprifuoco, alla chiusura delle scuole. L'Italia, però, è l'unico Paese che vuole limitare la libertà di spostamento tra Comuni vicini durante i giorni di festa. l'Italia è anche l'unico Paese dove nei giorni attorno al 25 dicembre si prevedono disposizioni più stringenti, mentre altrove si procederà con un allentamento per consentire alle famiglie di passare assieme il Natale. In Germania, durante il *lockdown*, si potranno incontrare al massimo cinque persone appartenenti a due diverse abitazioni, con l'estensione a dieci per i giorni dal 24 al 26. Anche in Austria il 24 e il 25 dicembre si possono riunire al massimo 10 persone, purché provenienti da un massimo di due abitazioni. In Svizzera è permessa la riunione di 10 persone fino al coprifuoco, che per il 24 e il 31 è portato all'una di notte. In Francia il coprifuoco è sospeso per la notte della vigilia. In Gran Bretagna, dove c'è il divieto di incontrarsi con persone non conviventi, gli appartenenti a tre diverse case tra il 23 e il 27 dicembre si potranno incontrare.

Questo approccio, che - come si vede - è quello comune europeo, dovrebbe assumere anche l'Italia per garantire alle famiglie di stare assieme a Natale. Per questo il Gruppo per le Autonomie non voterà né la mozione del centrodestra, che è troppo limitativa e fa riferimento solo al 25 dicembre, né quella della maggioranza, che dà al Governo la facoltà di rivalutare tutto, di cambiare di nuovo le carte in tavola, anche se tenendo conto della parità di trattamento tra Comuni piccoli e grandi. Per questo annuncio la nostra astensione.

colleghi, poco fa ascoltavo il collega del Partito Democratico che ci divideva tra aperturisti è una vecchia abitudine, quella degli amici di sinistra, di dividere il mondo tra parti, cioè il giusto e lo sbagliato, il bello e il brutto,

Responsabili sono coloro che prendono i provvedimenti, e cioè teoricamente il Parlamento, ma in pratica il Governo (fino a oggi è stato sempre così); innocenti sono i cittadini italiani che si trovano a essere soggetto di questi provvedimenti

teorico assolutamente parallelo, una sorta di *avatar* che governa una situazione drammatica e che sembra non stare alla realtà dei fatti? Noi siamo opposizione, colleghi, l'opposizione notoriamente non si fa carico delle azioni di Governo. L'opposizione denuncia, propone e, se condivide, partecipa alle decisioni. Questa volta abbiamo forzato la caratteristica del nostro ruolo e abbiamo suggerito, visto il provvedimento del 2 dicembre che conteneva restrizioni

alle condizioni di base della convivenza civile, alle nostre tradizioni, ai nostri momenti migliori: i giorni di Natale. Questo Questo è quello che teoricamente doveva fare la maggioranza. L'abbiamo fatto noi; ci siamo fatti carico di una mozione che addirittura proponeva degli elementi di soluzione, cosa che - ripeto - l'opposizione non è tenuta a fare. La mozione è stata faticosamente calendarizzata per oggi. Il presidente Conte ha dichiarato

Colleghi, voi avete deciso di abdicare in modo assolutamente scomposto. Noi ci prendiamo il merito di avervi aiutati a riportare nella sede opportuna questo dibattito. Voi continuate a cercare la soluzione migliore, che è lo scarico di responsabilità

nell'affrontare questa emergenza - colleghi, l'ho detto più volte - si è scelta sempre la strada certamente più facile, ma drammaticamente più

L'altra strada, quella che uno Stato serio e un Governo degno di questo nome con una sostanziale maggioranza avrebbero dovuto intraprendere, è quella del contenimento sanitario, collega Sileri,

Non abbiamo ancora i protocolli né delle domiciliari né della ospedalizzazione: un mare di inappropriatezza governa questa vicenda. Noi ancora non abbiamo visto, ammesso che esista, un piano vaccinale. Non parliamo del piano pandemico perché il tempo non mi aiuta - ne parleremo a tempo debito - ma un piano vaccinale, collega Sileri, lei l'ha visto? C'è? Basta che faccia cenno di sì o di un piano vaccinale. Il vostro supercommissario, generalissimo Arcuri scrive, un bando impegna quasi 600 milioni per individuare 3.000 medici e 12.000 infermieri; divide l'Italia in cinque zone e quant'altro. Dietro tutto questo c'è Arcuri che si crede Napoleone e si mette il cappello o c'è un piano vaccinale stabilisce chi fa che cosa, con quali dimensioni e con quali obiettivi di prevenzione e cura?

abbiamo esorbitato il nostro ruolo di opposizione e vi abbiamo suggerito una mozione che sostanzialmente diceva tre cose importanti:

proponeva di prevedere in ogni caso, nel rispetto del principio di precauzione e massima cautela, di consentire il ricongiungimento familiare con persone anziane, persone affette da disabilità o di figli con genitore separato. Esistono questi casi. Non si può fare di tutta l'erba

ai nostri operatori economici già drammaticamente falcidiati da questa epidemia. Rispetto a tutto ciò, abbiamo fatto la nostra parte. Voi,

in pompa magna sulla centralità del Parlamento e con Conte che dice addirittura "sotto la vostra responsabilità", con il ditino alzato come da tradizione familiare,

andrebbe affrontato a beneficio degli italiani che oggi, 16 dicembre, ancora non sanno che cosa dovranno fare fra nove giorni, il 25 dicembre?

Consentiamo lo spostamento dei nostri marinai che sono ancora in mano aun Paese straniero, affinché possano ricongiungersi con i loro familiari. Andiamoceli a prendere, come avrebbe fatto qualunque Stato degno di questo nome. Basta con questa vicenda scandalosa. Consentiamo almeno ai nostri marinai di passare il Natale con i loro cari. *(Applausi)*.

e cioè che la priorità, penso per tutti noi, e anche per i colleghi dell'opposizione, Non divido il mondo tra buoni e cattivi e, soprattutto, non mi metto mai a prescindere tra i buoni.

Ne parliamo troppo poco: qualcuno l'ha scritto ed io sono d'accordo, prima di tutto per le vittime, un numero spaventoso su cui dovremmo anche ragionare in un momento più serio,

che la discussione che stiamo facendo dovrebbe stare lontano dallo scontro politico. Del resto, abbiamo già avuto diverse riprove, colleghi: quante affermazioni sono state fatte, e dagli stessi modificate in modo radicale, proprio sul tema apri-chiudi, di più-di meno?

che, in una situazione così complessa, la risposta giusta in astratto non Certamente hanno ragione quelli che non assumono decisioni e hanno la possibilità di dire che la decisione assunta è sbagliata: si può fare anche questo gioco. Il collega Zaffini ha letto tante agenzie stampa e tanti comunicati e non ha letto uno - anzi ne ha letti due, ma gli consiglierei di leggere anche il terzo quale i Presidenti del Veneto e del Friuli-Venezia Giulia chiedono esattamente la zona rossa. Ma perché, colleghi? In In una riflessione sui dati che stanno emergendo sentono la responsabilità di evitare di

da una parte è nella Provincia di Ferrara e, dall'altra parte, è nella Provincia di Ravenna. Non c'è una soluzione che risolva tutti i problemi.

cogliamo nei provvedimenti fatti, compresi il decreto del 2 dicembre, il tema di conferire equilibrio alla questione dei piccoli Comuni, nella chiave di dare il più possibile la stessa equità

risarcimento. Voglio dire ciò che penso fino in fondo: voterò la mozione, ma voglio dire il mio pensiero.

dovremo dire con chiarezza quel che bisogna fare: dobbiamo stare a casa. Lo dico con grande serenità. Mi piacerebbe che su questo punto

Se qualcuno ha delle altre certezze, le espliciti - non cito il Presidente del Consiglio - naturalmente spiegando a tutti noi quale responsabilità è in grado di assumersi.

*(PD)*. Signor Presidente, autorevole Ministro, colleghi, il Partito Democratico ha posto con forza fin dall'emanazione dei recenti provvedimenti un tema che è emerso non per volontà di alcuno, ma perché,

che riterranno e con le indicazioni adeguate dal punto di vista tecnico-scientifico. Il punto che ci ha mosso

Sono battaglie che portiamo avanti all'interno del Partito Democratico, all'interno del Parlamento e nelle istituzioni italiane da tanti anni. Non possono esistere cittadini di serie A e cittadini di serie B. Non ci sono solo gli investimenti per i beni culturali dei grandi centri come accadeva tanti anni fa - credo che i Governi di centrosinistra abbiano determinato scelte diverse

ad esempio - nelle scuole, nei centri rurali, montani e isolani. C'è la necessità di investire in infrastrutture. C'è la necessità - e la pandemia lo ha dimostrato - anche di riconsiderare paradigmi e decisioni prese in passato, come sulla riduzione del numero degli ospedali e dei presidi sanitari. La salute è il principio che ci sta indirizzando nelle decisioni delle ultime ore e che ci deve anche insegnare che forse in passato qualche scelta è stata sbagliata.

seppure universale in termini generali, ipotizzava poi nell'applicazione specifica una differenziazione tra i cittadini: un cittadino di un piccolissimo Comune di cento, ma anche di mille abitanti, doveva rimanere all'interno di quel contesto territoriale, probabilmente senza servizi, soprattutto non poteva andare a fare visita al proprio genitore, a un parente di primo grado o a una persona molto vicina, a cui legato da un affetto Noi abbiamo chiesto di analizzare questa situazione, di verificarla e rimuoverla. Siamo contenti che il Governo abbia apprezzato questa istanza e ci stia lavorando, perché certamente il cittadino di quel piccolo paese di montagna o di campagna vivrebbe una situazione molto diversa da quella di un cittadino di una grande città,

importante che è stata accolta all'interno della mozione, ma non è certo l'unica. Ci rendiamo conto del quadro generale

del comitato tecnico-scientifico si possa operare. Qualora i dati, le indicazioni e le previsioni ci diranno che esiste il rischio concreto e gravissimo di un peggioramento della situazione, certamente siamo tra coloro i quali inviteranno il Governo a prendere i provvedimenti necessari, tenendo conto - com'è stato fatto per il decreto di inizio dicembre l'Italia è un Paese complesso, difficile, con territori diversi e situazioni regionali diverse. Io sono sempre sorpreso da alcuni toni delle opposizioni e del centrodestra: non sono d'accordo sulla mozione presentata; non sono d'accordo nell'identificare solo il giorno di Natale, nell'evidenziare il territorio provinciale. Io credo si debba fare tutti uno sforzo di grande responsabilità e comprensione della situazione. il migliore investimento, dal punto di vista economico e di prospettiva per il nostro Paese, è tornare a una situazione di normalità da un punto di vista sanitario. Essere i primi a uscire dalla crisi darà una spinta e un *boost* allo sviluppo, al recupero e alla capacità di rilancio del nostro sistema Paese. La sanità, la tutela della salute, il prendersi cura di ogni singolo cittadino sono i meccanismi che ci permetteranno, anche in chiave economica, di lavorare bene e di fare ciò che dobbiamo fare.

tutti questi operatori potranno lavorare anche durante le feste natalizie, ma, qualora non ci fossero le condizioni, bisogna essere che dobbiamo trovare le risorse economiche e finanziarie, con il decreto ristori cinque, per adottare i provvedimenti necessari e per ripristinare condizioni economiche sostenibili per chi vorrebbe fare libera impresa, ma oggi, vista la situazione sanitaria, non può. Signor Ministro, concludo dicendo che il Partito Democratico ha fatto presente delle istanze al Parlamento e al Governo apprezza la disponibilità dell'Esecutivo ad ascoltarle e ad intervenire, se riterrà, in maniera normativa o interpretativa sulla questione dei piccoli Comuni e degli spostamenti tra persone care, affinché possano incontrarsi anche nei giorni particolari che abbiamo davanti a noi. Chiediamo che si tenga conto del quadro generale, insieme al CTS, il Comitato tecnico scientifico, per assumere, eventualmente, ulteriori provvedimenti. Chiediamo che questi provvedimenti abbiano anche una logica legata al territorio, alla differente gravità e ai differenti numeri su tutto il territorio nazionale. Chiediamo anche un impegno preciso sui ristori, qualora qualche attività economica fosse ulteriormente penalizzata da decisioni che andremo ad assumere. La salute dei nostri concittadini, la salvaguardia della sanità pubblica e, in prospettiva, il rilancio economico e la salvezza del nostro Paese: queste sono le linee guida del Partito Democratico ed è per questo che votiamo favorevolmente a questa mozione.

Signor Presidente, colleghi, è con qualche imbarazzo che intervengo in dichiarazione di voto oggi.

In più, mi sento di dover fare più che una dichiarazione, una richiesta di voto alla maggioranza sulla nostra mozione, perché, dopo il parere del Governo, temo che la nostra mozione, come tanti nostri consigli e proposte, rischia di essere archiviata e questo non è un bene per il nostro Paese. orgoglioso del fatto che per primi noi abbiamo sollevato il problema e presentato una mozione unitaria del centrodestra. Da un lato, vorrei dire che è bene che la maggioranza abbia preso oggi coscienza del problema e, da quanto mi sembra di capire, si dia già per scontato il superamento dei limiti per il giorno di Natale. Questo limite lo dava già per superato, in modo meno brillante, il ministro Di Maio, che si è reso conto del problema, ma la risposta è stata assolutamente inadeguata se, oltre all'intervista che tutti abbiamo visto, ci dobbiamo rifare al *tweet* che ha lanciato, dicendo (sentenziando quasi): a Natale e a Capodanno permettiamo ai cittadini di spostarsi tra i piccoli Comuni. Questo sentenziare è di cattivo gusto e siamo tutti d'accordo nel ritenere assolutamente sgradevole, da parte di un Ministro, intervenire in questo modo e in questi termini. non ci voleva molto a capire che la Lombardia non è il Molise (10 milioni di abitanti non sono 300.000) e che Roma non è il paesino

Paese che, nel giro di 3, 4 o 5 chilometri vedono la presenza di 4 o 5 Comuni. Questo limite va superato con intelligenza e buon senso, il buon senso - purtroppo - sembra non appartenere a molte proposte che la maggioranza ha fatto in quest'Assemblea e al Paese.

- vogliamo frenare la pandemia, ma in troppe occasioni, come dicevo, ci si è dimenticati di usare il buon senso. Nessuno vuole un liberi tutti. Ma che senso ha aver chiesto ad alcune categorie costosissimi interventi per la messa in sicurezza delle loro attività, per poi decretarne la chiusura? Non ci si rende conto dei sacrifici che abbiamo chiesto a questi concittadini, ai dipendenti di queste attività? È vero, nessuno ha la certezza di quali misure siano davvero sufficienti.

ma, più semplicemente, tra buon senso e improvvisazione. *(Applausi)*. Noi assistiamo a una continua improvvisazione. ieri ne è stato l'esempio perché, al di là delle decisioni prese dalla Presidenza del Senato sulle inammissibilità, abbiamo approvato con un solo voto quattro rate di ristori. Questa è improvvisazione, non è programmazione; noi oggi abbiamo bisogno di programmazione, di serietà, di capacità messe in campo e di proposte che vengono fatte al Parlamento. Colleghi, è fondamentale - e questo è compito del Governo - trovare un equilibrio tra divieti, comportamenti virtuosi e vita necessaria, perché nella vita necessaria ci sono gli affetti e le relazioni, che durante le festività saranno anche limitabili, ma non sono eliminabili. Questo è il tema che oggi stiamo affrontando.

ma noi siamo per la libertà, che va coniugata con la responsabilità. Colleghi, non si devono chiedere ai cittadini sacrifici inutili e il rischio è che oggi noi continuiamo a chiedere sacrifici inutili, non utili; e questo non va bene. Nel frattempo tanti piccoli imprenditori - lo sapete anche voi - stanno rimettendo in gioco i propri beni personali nel tentativo di salvare le proprie imprese. non è sufficiente parlare - come fate nella vostra mozione - di ristoro proporzionale. Credo che, come da noi proposto e contenuto nella nostra mozione, si debba invece parlare di un vero risarcimento, che noi fissiamo almeno al 75 per cento. Guardate che, se non si interviene sostenendo le imprese, non si sostiene il lavoro. Più sostegno alle imprese vuol dire più lavoro per questo Paese e per i nostri cittadini. *(Applausi)*. La discussione di oggi in quest'Aula mi porta però alla

fatto bene a buttare la palla al Parlamento, perché è compito del Parlamento prendere alcune decisioni. Ma, colleghi, voi con la vostra mozione ributtate la palla clamorosamente e irresponsabilmente al Governo; e così non va. Perdonatemi, ma non è questa la centralità del Parlamento tanto evocata da tutti più volte in quest'Assemblea; non è questa la centralità del Parlamento. Per una volta che abbiamo la possibilità di decidere qualcosa e di dare una vera indicazione, noi rinunciamo?

servono più responsabilità, più buon senso, meno ottusità, meno casualità e improvvisazione. Noi continuiamo a lavorare per dare risposte agli italiani

Signor Presidente, colleghi, fortunatamente, essendo fra noi e non essendoci la diretta TV, possiamo ragionare ancora più tranquillamente di quanto non si possa fare di solito. Diciamoci alcune cose in totale serenità e poi continuiamo ad avanzare alcune proposte. Riparto dal collega di Forza Italia, che ha pienamente ragione. Da mesi

Poi, se uno decide, può decidere bene e può decidere per il meglio la volta dopo; però chiedere che scelgano altri non mi sembra responsabile da parte di nessuno di noi. Partiamo dai dati di fatto: quasi 66.000 morti. Questo è. L'Italia è il Paese col più alto numero di morti in Europa. Punto e a capo. Solo questo dovrebbe portarci a dire di lavorare insieme. È inaccettabile però se qualcosa va bene - e, ahimè, non sono tante le cose andate bene in questo periodo - è merito di chi sta al Governo, mentre, se qualcosa va male, è colpa delle opposizioni che sono irresponsabili, sovraniste, fasciste, antieuropeiste e negazioniste.

in un laboratorio cinese finanziato da alcune multinazionali senza alcun tipo di controllo *(Applausi)*, con l'Organizzazione mondiale della sanità che ha dormito, assente o complice, e mi domando perché i cittadini italiani continuino a finanziare un'organizzazione assente o complice. la Cina, da dove il contagio è partito, ovviamente per prima ha lavorato al vaccino e adesso sta vaccinando mezzo mondo dal Brasile al continente africano. Verrà il momento in cui quest'Aula, spero con responsabilità e unitariamente, chiederà un risarcimento danni, economici e morali, a coloro che hanno contagiato il resto del mondo

ha preannunciato 4 milioni di dosi entro gennaio: lo diciamo in quest'Aula oggi, 16 dicembre. Visto che fidarsi è bene e non fidarsi è meglio, vice ministro Sileri - lo abbiamo visto alla prova sulle mascherine, che non c'erano, abbiamo visto alla prova sulla riapertura delle scuole e abbiamo visto com'è andata a finire, lo stanno vedendo alla prova gli operai dell'Ilva - se arrivano i vaccini e non possiamo somministrarli perché mancano aghi e siringhe, facciamo il male del Paese. *(Applausi)*. È tutto sotto controllo?

dove, se qualcosa non funziona, non è colpa di chi governa, ma delle opposizioni. Avete stancato con questo ritornello, prendetevi le vostre responsabilità; il non ricordo non fa andare avanti un Paese.

«Signore e signori venghino, perché in Italia organizziamo la lotteria degli scontrini e chi va in un negozio entro il 31 dicembre vince un *bonus* da 150 euro». Poi si stupisce se la gente va in negozio a fare la lotteria dello scontrino. Ma mettiti d'accordo con te stesso: erano 13 giorni fa, 13 giorni fa e, dopo 13 giorni, il commerciante che ha speso 200 euro per aggiornare il suo macchinario, si accorge che il Governo lo chiude. Mettiamoci nei panni di un imprenditore o di un commerciante lombardo che è stato chiuso da ottobre da ottobre per scelta responsabile di Regione Lombardia e della comunità lombarda e che domenica scorsa è tornato in zona gialla, quindi a sorridere, a respirare e a passeggiare: adesso adesso lo rinchiudiamo in casa da questo venerdì? È semplicemente inaccettabile. *(Applausi)*. Il centrodestra prevede non regali o lotterie degli scontrini, ma un rimborso alla tedesca. Ci dite di fare come i tedeschi: facciamo come i tedeschi nelle chiusure, ma anche nei rimborsi - lo diceva una collega di Italia Viva - fino a 150.000 euro.

a nome ad esempio di quei commercianti fiorentini, che sono accampati e dormono giorno e notte in piazza a Firenze, che nel minuto in cui si annunciano eventuali nuove chiusure, vengano anche date disposizioni per bonificare, sui conti correnti, le migliaia di euro necessarie a queste persone per sopravvivere.

in quest'Aula non ho mai avuto modo di avere l'occasione di confrontarmi con uno dei protagonisti della situazione passata, presente e futura. Dalla

perché si è riaperto il sistema scolastico, che è la spina dorsale del Paese, con 8 milioni di studenti e un milione di insegnanti, senza aver fatto un "fico secco" sul trasporto pubblico locale e sull'affollamento nelle classi. Avete trattato i nostri bambini come cavie! Ora non vorremmo che il 7 gennaio si torni alla stessa storia e quindi chiediamo che nella manovra economica ci sia almeno un miliardo di euro per il potenziamento del trasporto pubblico locale. Potete chiudere tutti i negozi, i parrucchieri, gli estetisti, le palestre e le librerie a data da destinarsi, ma se piazzate migliaia di studenti negli autobus o in metropolitana, condannate a morte il Paese. *(Applausi)*. Occupatevi di scuola, di studenti, di classi e di insegnanti! una riflessione sul Natale. Non penso che in quest'Aula ci sia qualcuno che voglia malattia o morte: da questo punto di vista siamo tutti dalla stessa parte. Mi auguro che nessuno abbia in testa che qualcuno, per motivi politici, si auguri la morte o la malattia di nessuno.

quello che separa le famiglie il giorno di Natale sarebbe un dato solo italiano - secondo cui, chiudendo in casa mamme, papà, nonni, parenti, amici e nipoti il giorno di Natale, ci sarà un risultato positivo in termini di contrasto al virus? Non c'è, tant'è vero che in tutti gli altri Paesi europei, che hanno i nostri stessi problemi, si consente a cinque, sei, o al massimo 10 persone, di due o al massimo tre nuclei familiari, di trovarsi

si può trattare Roma come Taurianova, Pinzolo o uno dei borghi italiani, che non meritano discriminazioni. State discriminando gli italiani e le famiglie, tra italiani di serie A,

mi faccio 50 chilometri, cambio Provincia e vado a trovare mio figlio che vive con la sua mamma, da genitore separato, come ce ne sono milioni in Italia? Che rischio corro e che rischio faccio correre? Ditemelo. Che sia una giornata Che sia una giornata di buonsenso; prendetevi qualche responsabilità. Poi, è chiaro che molti colleghi di maggioranza, in queste ore, più che ai provvedimenti sulla salute, sul Natale, sul lavoro e sulla famiglia, hanno la testa al rimpasto, alla verifica, ai Servizi segreti. È triste che domani ci sia l'Italia appesa al confronto fra Conte e Renzi: non state dando un bello spettacolo della politica e della democrazia a questo Paese. Non è quello che gli italiani si aspettano in un momento così grave e delicato. Vi lasciamo ai vostri assembramenti di Governo e sotto Governo a Palazzo Chigi, e vi imploriamo di non rubare il Natale alle famiglie e ai bimbi di questo Paese che hanno già sofferto abbastanza. *(Applausi)*.

Signor Presidente, colleghi, stiamo vivendo un tempo straordinario, la più grande sfida dal Dopoguerra a oggi a difesa della salute umana. In pochi mesi abbiamo stanziato l'equivalente di tre manovre finanziarie. Questo Parlamento, nonostante le difficoltà, ha continuato a lavorare a provvedimenti che tutelassero le famiglie, le imprese e i lavoratori, mettendo al primo posto la vita dei cittadini. Oggi, alla luce dei dati, possiamo dire con certezza che il percorso è ancora lungo. Di questo nemico - che adesso gestiamo molto meglio - conosciamo ancora troppo poco, ma sappiamo con certezza che dovremo conviverci a lungo, continuando a scongiurare il rischio che il nostro Servizio sanitario nazionale collassi. Un Servizio sanitario nazionale vittima di tagli scellerati, perpetrati per decenni; un Servizio sanitario nazionale che ha retto solo grazie al sacrificio, anche fisico, dei nostri operatori sanitari. Viviamo una realtà diversa a cui non eravamo pronti; la nostra vita è condizionata da scelte forzate. Siamo tutti stanchi, ci manca ciò che eravamo prima, perché per la prima volta abbiamo visto limitati i nostri bisogni e i nostri diritti essenziali, quelli degli adulti e quelli dei bambini. Vedere i nostri ragazzi isolati dai propri amici, gli anziani lontani dai familiari, i disabili senza il supporto degli operatori che li accompagnano è straziante, ma abbiamo capito che isolamento non vuol dire solitudine e che il distanziamento sociale rappresenta un gesto d'amore verso i più fragili. Siamo ormai a più di 71 milioni di casi confermati nel mondo, più di 1,5 milioni di morti, più di 65.000 morti solo in Italia, e molte delle persone decedute erano soggetti fragili, soprattutto anziani: la memoria storica di un Paese, coloro che hanno contribuito a fondare il mondo in cui viviamo. Abbiamo operato, per la prima volta nella storia, prendendo delle decisioni seguendo il metodo scientifico; eppure, oggi, in quest'Aula, discutiamo se alleggerire o meno le restrizioni previste dall'ultimo DPCM. Certo, abbiamo tutti bisogno di un po' di leggerezza; vogliamo intravedere la fine di questo incubo e vorremmo tutti poter dire ai cittadini che il peggio è passato. Purtroppo, però, i dati del monitoraggio dei contagi, diffusi dall'Istituto superiore di sanità e ripresi dal comitato tecnico-scientifico, confermano la necessità di mantenere in vigore le restrizioni attualmente in atto. Secondo gli scienziati, per la prima volta nella seconda ondata, la velocità di trasmissione dell'epidemia in Italia sta rallentando, e l'incidenza a livello nazionale sta diminuendo. Tuttavia questo dato si accompagna ad un lieve aumento delle ospedalizzazioni in area medica e in terapia intensiva e a un'incidenza ancora troppo elevata, con circa 700.000 persone attualmente positive, una mole che rende impossibile il tracciamento, anche con un numero tre volte maggiore di test, senatore Zaffini. Se è vero che comunque le misure restrittive sono riuscite ad allentare la pressione sugli ospedali e sulle terapie intensive, il dato di occupazione dei pazienti Covid nei reparti continua ad essere superiore al 40 per cento e nelle terapie intensive al 30 per cento in ben 15 Regioni. Ciò significa che siamo ancora oltre la soglia critica e non possiamo non usare cautela. Inoltre, dobbiamo considerare che i dati riportati oggi si riferiscono a due settimane fa e se in questi giorni di riaperture stanno aumentando i casi, perché sono aumentati i contatti e gli spostamenti, lo sapremo solo tra un po'. Dobbiamo anche tener presente che diversi *report,* tra cui quello della Fondazione Gimbe, ci mettono in guardia sull'arrivo di una tempesta perfetta, causata dall'avvento dei mesi invernali, dall'imprevedibile impatto dell'influenza stagionale, dal legittimo entusiasmo per il vaccino in arrivo, che potrebbe spingerci ad allentare le misure restrittive e portarci verso una terza ondata di contagi. In questi mesi abbiamo più che raddoppiato i posti in terapia intensiva e subintensiva, abbiamo cercato di garantire ad ogni paziente un trattamento rispettoso della dignità umana, grazie al sacrificio e alla resilienza di tutto il nostro personale sanitario Non siamo però riusciti ad alleviare la pressione costante sui nostri ospedali, indeboliti da decenni di tagli. In questi mesi, grazie alla disciplina, alla pazienza e alla responsabilità dei cittadini italiani, siamo riusciti a tenere sotto controllo la curva dei contagi, abbiamo guadagnato tempo e questo tempo prezioso va certamente utilizzato per rafforzare concretamente il nostro Servizio sanitario nazionale attraverso una collaborazione più efficace tra Stato e Regioni, che devono mettere in atto immediatamente le direttive ministeriali di riorganizzazione della rete ospedaliera e territoriale. Il senatore Zaffini e anche il senatore Salvini parlavano di scelta di voler abdicare, di non voler decidere. Invece noi ancora una volta oggi prendiamo delle decisioni politiche, che non devono prescindere dall'evidenza scientifica Sono decisioni sofferte, altro che strada più semplice, ma decisioni necessarie perché non serve affidarsi alla speranza, ma seguire il metodo scientifico. Questo percorso che ci porta fuori dall'emergenza non è una corsa ai cento metri, ma una maratona. Grazie alla scienza in questi mesi abbiamo messo a punto protocolli per limitare la sintomatologia e i danni da Covid, sono stati testati farmaci antivirali e anticorpi monoclonali; siamo nelle fasi finali di approvazione di diversi vaccini che saranno gratuiti e disponibili per tutti, un traguardo straordinario mai raggiunto prima Al senatore Paroli, che parlava di improvvisazione, di incertezza sulle misure da prendere, al senatore Salvini, che ancora parla di virus creato in laboratorio, di assenza di evidenza scientifica, dico che proprio in questi giorni la scienza, attraverso un bellissimo lavoro di metanalisi pubblicato sulla ha dimostrato che, tra tutte le misure non farmacologiche messe in atto dai Governi di tutto il mondo, valutando più di 6.000 parametri in 79 luoghi diversi, usando quattro approcci statistici, nessun intervento riesce da solo a portare l'indice di trasmissibilità (il cosiddetto indice RT) a meno di uno e i dati riportati in questo importante studio dicono che le misure più efficaci per allentare e ridurre la diffusione del virus nella popolazione si sono dimostrati essere proprio le chiusure dei luoghi in cui le persone si assembrano in piccoli o grandi gruppi, quindi i luoghi di aggregazione sociale ma anche le riunioni familiari sembrano essere i principali fattori di rischio in questa pandemia. questo che nella mozione di maggioranza che il MoVimento 5 Stelle appoggia ribadiamo che, in attuazione del principio di massima precauzione e della necessità di tutelare la salute dei cittadini, l'adozione di qualsiasi misura sia in senso restrittivo che ampliativo deve essere valutata sulle evidenze scientifiche relative all'andamento della curva epidemiologica, garantendo la massima equità di trattamento tra i cittadini residenti in Comuni di diverse dimensioni e prevedendo, nell'eventualità di nuove restrizioni, misure di ristoro economico e questo punto sui ristori è stato aggiunto nella mozione di minoranza solo dopo aver letto il nostro testo.

quel senso di appartenenza a una comunità che solo se unita può uscire più forte di prima da questa esperienza tragica. Se saremo in grado di non cedere alla tentazione dei numeri incoraggianti, allora riusciremo a tutelare al contempo la salute, l'economia e la vita sociale, mettendo in sicurezza il nostro sistema sanitario. Non dobbiamo tornare alla normalità pre-pandemia, dove per normalità si intendeva un Paese che non destinava sufficienti risorse alla sanità e alla scuola, un Paese in grave ritardo nella digitalizzazione e nella promozione della sensibilità ambientale, ma dobbiamo costruire una nuova normalità e immaginare un nuovo modello di società che non lasci indietro nessuno e che sia capace di generare bene e non solo di consumare bene, che produca cose che abbiano un valore e non solo un prezzo, e noi, in quest'Aula, abbiamo la responsabilità di coltivare la memoria, anche quella recente di ciò che stiamo vivendo in questi mesi, non solo facendo fronte all'emergenza, ma con il compito più impegnativo di generare il futuro, non di attenderlo per essere all'altezza della storia e saper incarnare e realizzare i sogni e la visione di questo meraviglioso Paese.

devo ammettere che in quest'Aula ho sentito parlare di cose che forse è veramente meglio che decidano il Governo e il Ministero della sanità e non noi.

la mia voce roca è veramente insopportabile. Siete veramente dei maleducati quando fate così.

Molti piccoli Comuni delle mie vallate sono praticamente tutti infetti. Favorire lo spostamento, in questi giorni, tra piccoli Comuni, tra Regioni...

una possibilità di movimento e di incontro in nome di un'identità culturale, affettiva e quant'altro, danneggerà gli italiani. Sarebbe servito un *lockdown* secco

che si facciano sberleffi, applausi e grida, quando si tratta un argomento così importante *(Commenti)*, soprattutto sulla mia persona, visto che ho sempre rispettato in silenzio il parere di tutti.

una nuova finestra"). L'ordine del giorno reca la discussione congiunta dei documenti VIII, nn. 5 (Rendiconto delle entrate e delle spese del Senato per l'anno finanziario 2019)

*relatore*. Signor Presidente, come ogni anno l'Assemblea del Senato si trova ad esaminare gli atti relativi al bilancio interno dell'Istituzione. Questa volta si tratta del rendiconto delle entrate e delle spese del Senato per l'anno finanziario 2019 e del progetto di bilancio relativo all'anno 2020, che il Consiglio di Presidenza ha deliberato nella riunione dello scorso 24 novembre. Limitandomi a un esame essenziale di questi due documenti contabili e iniziando dal rendiconto relativo allo scorso esercizio finanziario, osservo innanzitutto come la spesa complessiva effettiva (al netto dei risparmi da versare allo Stato) sia risultata pari, nel 2019, a euro 486.342.227,17 in in diminuzione di oltre 760.000 euro rispetto al dato consuntivo dell'esercizio 2018 e addirittura di circa 34 milioni di euro rispetto al dato consuntivo dell'esercizio 2012. Va inoltre considerato che questo dato di riduzione della spesa, essendo espresso in termini nominali, non tiene conto della dinamica inflazionistica e dunque risulterebbe ancora più marcato, ove venisse espresso in termini reali. Peraltro, le entrate del Senato evidenziano che la dotazione finanziaria è rimasta invariata dal 2012 nella misura di circa 505 milioni di euro. Per conseguenza, rispetto

anche nell'esercizio 2020 - così come si può evincere dal bilancio di previsione per l'esercizio in corso - la riduzione cumulata dall'inizio della scorsa legislatura risulta pari addirittura a 172,8 milioni di euro. La costante riduzione della spesa negli ultimi anni si è dunque accompagnata a una sostanziale stabilità della principale entrata del Senato, con assestamento però di quest'ultima su un livello significativamente più basso rispetto agli anni antecedenti alla crisi del 2011. Per quanto riguarda la composizione della spesa, quella di funzionamento è risultata pari, nel 2019, al 55,4 per cento della spesa complessiva, contro il 44,6 di quella previdenziale, con un leggero decremento rispetto al 2018 della quota destinata al funzionamento dell'Istituzione e alle spese in conto capitale. Per quello che riguarda il bilancio di previsione 2020, oltre al dato già evidenziato della minor dotazione richiesta anche per l'anno in corso, si registra, per quanto riguarda le spese di natura previdenziale, una variazione di poco superiore all'1 per cento rispetto al 2019. Tuttavia, va rilevato che tale importo comprende anche le somme accantonate a seguito delle riduzioni introdotte sia per i vitalizi sia per i trattamenti pensionistici. In particolare, si evidenzia che i risparmi dovuti all'applicazione della riforma del calcolo dei vitalizi, approvata nel corso dell'anno 2018, sono stati lasciati in un apposito fondo, istituito prudenzialmente fino alla fine dell'*iter* processuale in corso presso gli organi di giustizia interna. Anche per quanto concerne l'applicazione del comma 261 della legge n. 145 del 2018, che prevede la riduzione dei trattamenti pensionistici superiori a determinati importi annui lordi, si è proceduto all'istituzione del «Fondo risparmio sui trattamenti pensionistici di importo elevato», così come stabilito dalla stessa legge, al comma 265. Occorre evidenziare, inoltre, la circostanza che, nello scorso esercizio finanziario, la spesa corrente obbligatoria ha rappresentato ben il 91,18 per cento di tutte le spese del Senato, anche se, a partire dal 2016, si è registrata una lieve tendenza alla riduzione di questo aggregato, che comprende i risparmi e i costi per senatori ed *ex* senatori, personale di ruolo, in quiescenza o estraneo all'Amministrazione, nonché tutti gli oneri collegati, quali quelli fiscali e previdenziali. Si registra altresì una leggera diminuzione, nel triennio 2017-2019, anche per quanto riguarda la spesa corrente di funzionamento in senso stretto, un aggregato che si compone di tutte le spese sostenute per l'erogazione di servizi e forniture di supporto al funzionamento del Senato, quali le prestazioni professionali per l'Amministrazione, le spese per l'attività delle Commissioni, i costi per i servizi informatici, di comunicazione, assicurativi, di ristorazione, di trasporto, di locazione, delle pulizie ed altri. Viceversa, Viceversa, risulta in aumento la spesa in conto capitale, che tra il 2017 e il 2019 è passata da 1.702.323,23 euro a 2.066.679,44 euro, anche se nel 2018 era risultata più alta di circa 400.000 euro rispetto a quella registrata nel rendiconto 2019. La spesa in conto capitale, che costituisce l'aggregato meno rilevante in termini assoluti tra quelli precedentemente citati, comprende le spese per l'acquisto di beni mobili inventariati, le spese di manutenzione straordinaria, nonché quelle di acquisto e conservazione del patrimonio della Biblioteca e dell'Archivio storico. A fronte di una così marcata riduzione delle spese come quella registrata a partire dal 2012, la sfida, naturalmente, è stata ed è tuttora quella di rendere compatibili i risultati finanziari conseguiti, che testimoniano la partecipazione del Senato allo sforzo di stabilizzazione della finanza pubblica compiuto negli ultimi anni, con il mantenimento di un elevato *standard* qualitativo dei servizi erogati, tanto più in un contesto che ha visto, almeno fino alla fine del 2019, una costante riduzione del personale di ruolo dell'Amministrazione. PRESIDENTE. Ha

Presidente, onorevoli colleghi, anche a nome dei colleghi Questori, Bottici e Arrigoni, sottopongo oggi pomeriggio all'attenzione dell'Assemblea il rendiconto delle entrate e delle spese del Senato per l'anno finanziario 2019 e il progetto di bilancio interno del Senato stesso. Nell'attuale contesto di emergenza del Covid-19, che sta avendo un impatto drammatico su tutto il Paese, a livello sia sanitario sia socio-economico, mi preme sottolineare le valutazioni che abbiamo fatto in questi mesi per quanto riguarda il Senato stesso. Sono ben consapevole che si tratta di misure di carattere generale di tipo sanitario-organizzativo e di disciplina del lavoro che voi, cari colleghi, ben conoscete, ma che, ancora una volta, è importante ribadire. Sin da subito abbiamo messo in atto tutta una serie di atti e indicazioni, da un punto di vista sanitario-organizzativo, per far fronte a questa epidemia. importanti, sentiti i servizi di competenza e di protezione e il medico competente, in modo particolare il Direttore del Polo sanitario, dottor Marini, che vorrei qui in premessa ringraziare per il lavoro che ha fatto tutto insieme

ci siamo dati sono la sicurezza sanitaria (quindi la tutela della salute come fattore fondamentale e prioritario) e la continuità dell'attività legislativa dell'organo costituzionale del Senato. Abbiamo adottato tutta una serie di misure di carattere generale e sanitario e siamo intervenuti con una serie di disposizioni sul lavoro, in modo particolare con lo *smart working* per tutti i nostri dipendenti e collaboratori. Siamo intervenuti con il documento sui rischi biologici da contagio, a integrazione del misure di carattere organizzativo. Abbiamo garantito che l'attività legislativa e l'esame degli importanti provvedimenti legati all'emergenza procedessero con la partecipazione attiva di tutti noi senatori, assicurando il rispetto di tutte le norme

- delle Commissioni e delle Giunte. Da ultimo, proprio per dare un'ulteriore garanzia rispetto all'andamento dell'epidemia, il Collegio dei Questori ha dei Questori ha ritenuto opportuno richiedere un parere per la valutazione del rischio di trasmissione di microrganismi in aria nell'Aula legislativa e nelle Commissioni. Proprio per questo, come sapete,

Negli ultimi anni - dal 2012 al 2018 - abbiamo avuto un *trend* di diminuzione pari a 34 milioni di euro. Credo che questo sia un aspetto fondamentale e importante. Abbiamo avuto inoltre una riduzione della spesa del Senato rispetto a quella dello Stato, passando allo 0,056 per cento. Credo che questa sia un'attenzione che, come Questori e come organo del Senato, abbiamo sempre messo in atto per dare una risposta concreta, tra l'altro di quest'anno (ma non solo) di grande crisi economica per le nostre famiglie. Credo che questo sia uno degli altri aspetti altrettanto importanti. Il rendiconto prevede di accertare un avanzo di esercizio per l'anno finanziario 2019 pari a 61,15 Sono risparmi importanti, dovuti a una gestione accorta e oculata del livello amministrativo. Altrettanto vale per il bilancio dell'assistenza sanitaria dei senatori, che - come voi sapete - è totalmente

abbiamo dovuto fare tutta una serie di interventi altrettanto fondamentali e importanti. Continuiamo con la richiesta di una minor dotazione di 21,6 milioni all'anno, che ha portato in questi ultimi anni a ultimi anni a un minor impatto sulla finanza pubblica di 173 milioni di euro circa. Credo che questo sia un altro degli aspetti importanti, assieme

che ci ha portato ad avere 116 milioni di risparmi. Credo che questo sia una uno degli aspetti, altrettanto importanti, che vedono tutta una serie di operazioni fatte, a cominciare dalle integrazioni funzionali delle amministrazioni di Camera e Senato. Stiamo portando avanti insieme tutta una serie di procedure per avere il miglior risparmio e il miglior prodotto rispetto al mercato; credo che questo sia uno degli aspetti importanti. Vorrei ricordare inoltre a quest'Assemblea che tutte le procedure di gara sono gestite in via interamente elettronica mediante l'utilizzo di una piattaforma

Anche su questi aspetti abbiamo una serie di risparmi e altrettanto vale per quanto concerne le indennità parlamentari e le competenze accessorie, con un'ulteriore diminuzione che vorrei citare: dal 2001 al 2020 si è passati circa dal 19 al 10 per cento, praticamente dimezzando i costi delle indennità stesse. Il Senato della Repubblica - forse questa è una cosa strana agli occhi dei cittadini e di ognuno di noi

Credo che siamo al di sotto di tutte le medie europee, in senso positivo; paghiamo praticamente in pochissimi giorni. È un dato del 2019, ma,

la nostra la nostra amministrazione nel suo contesto generale. Fondamentale è dunque l'aspetto delle risorse umane. Come sapete, siamo sotto organico in maniera importante.

uno dei temi che nel 2021 dovremo riprendere con forza, per dare la possibilità a tutti i nostri uffici e all'amministrazione stessa di lavorare nel migliore dei modi e in maniera efficiente.

dei collaboratori parlamentari. Abbiamo avviato un tavolo di confronto con i colleghi della Camera dei deputati che riguarda lo *status* dei collaboratori parlamentari, nell'intento di trovare una soluzione condivisa sull'argomento. La questione

del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Ogni senatore può chiedere quindi l'accredito presso il Senato della Repubblica esclusivamente per i collaboratori con i quali abbia instaurato un rapporto di lavoro di durata non inferiore a sei mesi, a titolo oneroso, consegnando al Servizio di questura e del cerimoniale copia della comunicazione del contratto. Con una delibera che è stata fatta a suo tempo, nella regolamentazione della figura dei collaboratori parlamentari è stata definita una prestazione minima di venticinque ore mensili,

Come ho già detto prima, però, ribadisco l'importanza di un tavolo di confronto con l'altro ramo del Parlamento, proprio al fine di definire soluzioni condivise e individuare così una risposta concreta alla questione dei

essere valido. Andando oltre, abbiamo fatto tutta una serie di politiche *green* all'interno del Senato. Stiamo lavorando sull'efficientamento energetico e sulla riqualificazione delle aree adiacenti ai palazzi. Si sta realizzando un piano per il superamento delle barriere architettoniche. Questi

digitale per la presentazione informatizzata degli atti parlamentari, come ad esempio gli emendamenti, anche mediante firma elettronica, da parte sia dei Gruppi parlamentari che di tutti i senatori. Quindi informatizziamo e andiamo

interventi, realizzati proprio per dare la miglior possibilità di lavoro ai nostri colleghi. Certamente c'è sempre tanto da fare e credo sia importante evidenziarlo, ma, anche in un momento di grande difficoltà, credo che siamo riusciti a superare tantissimi problemi. Mi avvio alla conclusione,

con la speranza che effettivamente si avvii un percorso, che possa portare a una maggiore trasparenza, che ci è richiesta dalla popolazione, sui contratti dei nostri collaboratori, che spesso e volentieri purtroppo, sono effettivamente oggetto di distorsioni e di irregolarità.

per la razionalizzazione delle spese del Senato, ma soprattutto della qualità delle stesse, nel rispetto del principio certamente dell'economicità, ma anche dell'efficienza. La nostra è, infatti, un'istituzione che ha bisogno di funzionare al meglio per le competenze che ci vengono assegnate. Sto pensando, per esempio, all'importanza di aver sbloccato il *turnover* e di aver avviato un processo di nuove assunzioni, anche se i concorsi in questo momento sono sospesi per l'emergenza sanitaria. Partendo dal rendiconto delle entrate, vorrei evidenziare che, a fronte di una dotazione finanziaria invariata intorno ai 505 milioni di euro, le spese effettive sono pari a 486,342 milioni di euro, in leggera diminuzione rispetto al dato del 2018.

così come rispetto alla spesa corrente obbligatoria che - ricordiamolo - copre il 91 per cento di tutte le spese del Senato e si suddivide nella spesa per senatori ed ex senatori, Gruppi parlamentari, ma anche personale dipendente in servizio e in quiescenza, così come gli oneri previdenziali e fiscali a carico dell'amministrazione. Parliamo di un risparmio importante, visto che nel bilancio 2018 avevamo registrato 441,985 milioni nel bilancio 2019, invece, attestiamo la spesa a 413 milioni di euro. Un risparmio significativo, così come per quanto riguarda le spese per servizi e forniture. Vorrei ricordare le principali spese in conto capitale che sono già state evidenziate in parte dal questore De Poli, le spese che abbiamo sostenuto per i lavori di riqualificazione dei palazzi del Senato, quali, per esempio, per Palazzo Madama, il nuovo sistema video dell'Aula e il il rifacimento della 2a Commissione al piano ammezzato; quindi, spese importanti di manutenzione straordinaria. Un percorso che continua con il bilancio di previsione per l'anno 2020, redatto secondo le regole di contabilità generale, ma anche le regole interne proprie del Senato, che evidenzia e conferma l'obiettivo del risparmio della spesa ad oltre 700.000 euro rispetto allo stesso dato del 2018. Un risparmio che, in otto anni - questo mi preme sottolinearlo - quindi dal 2013, si attesta a 288 milioni di euro; quindi, una riduzione del peso finanziario del Senato sulla finanza pubblica, con

per la riduzione dei trattamenti pensionistici superiori a determinati importi, che quindi va a costituire uno specifico fondo di risparmio; l'altro l'altro riguardante le spese di natura previdenziale, in applicazione della riforma del 2018 per la riduzione dei vitalizi: un fondo istituito in maniera prudenziale-precauzionale, in attesa che termini l'*iter* processuale interno agli organi di giustizia. Mi sembra anche questa una scelta intelligente nella gestione finanziaria. Come dicevamo prima, c'è stata una riduzione importante per quanto riguarda l'importo complessivo della massa stipendiale, notevolmente ridotto in otto anni, dal 2012, del meno 22 Aggiungo infine che, oltre ai princìpi di economicità e di qualità della spesa, va anche sottolineato l'impegno per una maggiore trasparenza della gestione finanziaria, fino alla pubblicazione dei conti riguardanti i Gruppi parlamentari non solo sul sito, ma proprio in allegato ai provvedimenti in esame. Mi sembra che anche questa scelta sia da evidenziare. Vorrei fare una sola osservazione, che si provveda cioè quanto prima, grazie allo sblocco del *turnover,* a fornire i nostri uffici del personale in modo adeguato e sufficiente a poter garantire una lineare attività per l'esercizio delle funzioni che ci sono assegnate e quindi per dare il massimo dell'autorevolezza ai compiti che questo Senato è chiamato a svolgere.

Fatemi dire che credo sia giusto replicare un ringraziamento non retorico ma sentito a chi, come il dottor Marini, ha avuto e ha tuttora la responsabilità di guidare il presidio sanitario di questa Istituzione ma anche la lungimiranza di mettere in campo un meccanismo di prevenzione con l'obiettivo di mettere in sicurezza i parlamentari e i loro collaboratori, ma soprattutto tutti coloro che questi Palazzi li frequentano, li abitano e li vivono quotidianamente, anche quando sembrava che un certo suggerimento in relazione ai sistemi di protezione fosse quasi sciamanesimo, come se quella pandemia che poi a un certo punto ci ha colpito disastrosamente non non fosse alle porte, come poi è accaduto. Di questo elemento di lungimiranza dobbiamo dare atto al dottor Marini, naturalmente in un rapporto molto stretto con il Consiglio di Presidenza e con il Collegio dei Senatori Questori che ha avuto

mia percezione, anche in presa diretta essendo membro del Consiglio di Presidenza, è quella di un lavoro condotto in ragione

valorizzato in un momento in cui evidentemente, anche nel rapporto con l'opinione pubblica, fare operazioni di questo genere non è mai semplice, perché non si sa mai qual è la linea

a tutti i colleghi. Sono molto contento di questa assunzione, nella relazione del senatore De Poli, di un tema importante come quello dell'inquadramento dei collaboratori parlamentari sul piano della loro professione e professionalità.

alle prese con la possibilità di depositarli e non lo ha fatto proprio perché l'orientamento di fondo è quello di costruire un passaggio all'insegna

vanno bene gli impegni assunti. Bisogna prendersi la responsabilità di legare alcuni ragionamenti che spesso echeggiano in quest'Aula, e che sono anche oggetto di una traduzione in termini di iniziativa legislativa che spesso esercitiamo, con i comportamenti che poi mettiamo in campo e con la coerenza di quei comportamenti. Spesso, infatti, parliamo della dignità del lavoro, di come - tanto più nella fase che stiamo vivendo - dobbiamo aggredire il tema della precarietà del lavoro e di chi questa precarietà la vive quotidianamente, quindi coerenza vorrebbe che questo ragionamento venisse legato, nel caso specifico dei collaboratori parlamentari, ad un impegno diretto a un inquadramento professionale. Ci sono dei modelli che non dobbiamo inventarci - penso al modello europeo inteso innanzitutto come quel modello a cui fa riferimento il Parlamento europeo - che si possono implementare con grande semplicità, nel segno della trasparenza, del rispetto e della dignità di chi lavora con noi e penso sia un modo per

casta che ha interesse a opacizzare qualsiasi ragionamento. Possiamo dare un contributo ulteriore a uscire da questa ombra opaca proprio facendo un'operazione positiva per i collaboratori parlamentari ma anche per noi, nel senso di rendere la nostra attività ancora più efficace, più funzionale e soprattutto più disponibile a costruire un legame tra quello che facciamo e la vita reale delle persone.

compiuto in questi anni, che è andato nella direzione di razionalizzare molti costi e di rendere più moderna questa Istituzione. Istituzione. Non li ripeterò, ma un'occasione come questa ci può essere utile anche per fare qualche ragionamento che va verso il futuro. il futuro. Se mentre i costituzionalisti e anche molti di noi si interrogavano sul voto a distanza qui si è lavorato e si è continuato a svolgere le funzioni fondamentali per il Paese e per la sua democrazia credo sia stato grazie alla capacità organizzativa del Senato, di tutti i suoi dipendenti, dei funzionari dirigenti e del Collegio dei Senatori Questori, che hanno organizzato il lavoro e di questo bisogna dare atto. *(Applausi)*. La discussione è ancora in corso sul tema del voto a distanza e quindi questo è un elemento di modernizzazione delle istituzioni che dobbiamo ma nel frattempo noi siamo qui e credo che questo sia un fatto da sottolineare. Il discorso che ha fatto il senatore De Poli è importante, è stato un riassunto decisivo: questo è stato un anno complicato e complesso,

molto velocemente, ma con capacità professionale e con la sicurezza sanitaria garantita dallo *staff* del dottor Marini, attraverso un insieme di decisioni che dal segretario generale, dottoressa Serafin, ai vice segretari Toniato e Sandomenico, e ovviamente al Consiglio di Presidenza, al Consiglio di Presidenza, hanno dato esiti importanti dal punto di vista dell'efficacia. Abbiamo davanti un futuro, che ormai è alle porte, che prevede la riduzione del numero dei parlamentari. se immaginassimo che il *trend* che abbiamo impostato in Senato in questi anni per la gestione del bilancio non sia influenzato da questa modifica costituzionale, credo che faremmo un errore clamoroso. Il bilancio del Senato, infatti, è strettamente collegato alle scelte organizzative che riterremo essere adeguate e necessarie per rifunzionalizzare l'Istituzione rispetto ai nuovi numeri e alle nuove necessità. Quindi è un tema di modernizzazione, di digitalizzazione, ma anche di organizzazione del lavoro dei senatori e dei Gruppi politici. È un lavoro che è partito con la revisione dei Regolamenti

per garantire la rappresentanza democratica nel nostro Paese all'interno di questa Istituzione. Saranno meno persone, ma la loro capacità di lavoro e di rappresentare il territorio dal quale provengono deve essere intatta, anzi, deve potenziata e supportata in misura maggiore proprio perché ci sarà una diversa ripartizione dei carichi di lavoro e delle responsabilità che dovranno prendere carico. Questo è un anno di svolta, di progettazione, di programmazione sia dal punto di vista dei Regolamenti che dal punto di vista del bilancio. Il tema degli assistenti parlamentari è centrale rispetto a questo

prima di tutto si debbano definire le strategie e poi l'organizzazione dovrà essere capace di accompagnarle in modo efficace. Abbiamo anche un'altra possibilità storica. possibilità storica. La riforma riguarda Camera e Senato. La necessità di intervenire sui Regolamenti e sull'organizzazione non è solamente nostra, è anche dell'altra Camera, quindi abbiamo un'occasione di coordinamento ancora maggiore rispetto a ciò che è stato tentato negli anni passati. del fatto che nella quotidianità della vita del Senato si nota la capacità dell'Istituzione e di tutti i suoi uffici di mandare avanti con progressività i lavori di ristrutturazione, i lavori di ammodernamento tecnologico, di superamento delle barriere, di efficientamento energetico, con l'attenzione alla sostenibilità che anche questa Istituzione ha messo in campo nella gestione del ciclo dei rifiuti all'interno dei Palazzi. Ci sono altri temi da trattare, relativi, ad esempio, al lavoro a distanza perché una quota del lavoro che facciamo può essere sviluppato - e lo abbiamo visto in questi mesi - attraverso questa modalità, ma c'è anche un tema di *cybersecurity* che io non sottovaluterei rispetto alla ancora tutti per il lavoro che avete svolto. Ovviamente il nostro voto sarà favorevole.

l'immagine del Senato che è emersa dalla descrizione di questo bilancio è sommamente virtuosa sotto tanti punti di vista, Il primo è che tra i tre senatori Questori, che rappresentano anime diverse del Senato, sembra proprio che ci sia un grande affiatamento, una grande capacità di collaborazione, al di là di spaccature ideologiche o di prevaricazione. Questa quindi è la dimostrazione che si può lavorare insieme e che la collaborazione è possibile anche nella diversità delle provenienze politiche. Un'altra immagine positiva che viene fuori dalla descrizione che è stata fatta è quella di un Senato che, davanti a un'emergenza sociale come quella che stiamo vivendo, davanti a un livello di impoverimento generale del Paese, è stato capace di risparmiare e di farlo su tutte le voci del bilancio: ha risparmiato sulle quote del personale, sulle quote del trasferimento ai senatori delle loro competenze parlamentari parlamentari e, complessivamente, nella gestione dei servizi. È quindi un Senato consapevole della sua responsabilità sociale d'impresa, chiamiamola così. così. L'altro aspetto che è venuto fuori con grande attenzione è la sensibilità alla dimensione tecnologica avanzata del Senato, e molti sono gli esempi che si possono fare in questo caso e che sono stati anche fatti. A me interessa sottolineare che questo è un Senato capace di pensare tecnologicamente e di tradurre le possibilità che la scienza e la tecnica mettono a nostra disposizione in soluzioni operative immediatamente efficaci per tutti. È stata citata prima anche dal collega Collina la possibilità del lavoro in *smart working*, la possibilità del voto anche a distanza attraverso i *tablet*, la possibilità che abbiamo sperimentato tutti in questo periodo di organizzare *webinar* di altissimo profilo tecnologico, con una qualità di immagine e di audio e una sicurezza nei collegamenti che veramente fa invidia rispetto a situazioni analoghe che abbiamo sperimentato. un Senato capace di pensare anche in termini forti di prevenzione e di tutela della salute. Tutti noi abbiamo potuto fare tutti i tamponi che abbiamo voluto: ogni volta che il dubbio si è insinuato in qualcuno di noi di aver potuto essere esposti al contagio, siamo potuti andare a bussare alla porta del già pluricitato dottor Marini e abbiamo non solo trovato sempre ascolto, ma anche soluzioni che arrivavano prima, più e meglio. Penso anche all'operazione delle vaccinazioni: tutti quelli di noi che hanno voluto vaccinarsi dal virus dell'influenza, hanno potuto farlo e non hanno trovato resistenza di nessun tipo. Ora mi chiedo: un Senato così virtuoso perché diamine in altri momenti della sua vita deve essere scavalcato a destra o a sinistra da altre strutture? Perché deve essere svuotato di senso nella sua funzione più profonda, quella che definisce proprio il *core* del Senato, che è, ad esempio, la sua capacità normativa la sua capacità normativa e di prevenzione? Se penso al caos di ieri sera, attraverso i famosi decreti-legge ristori, penso che se il Senato avesse potuto lavorare, avrebbe lavorato con questo senso dell'economia, con questo senso dell'efficienza, con questo senso di interesse per il bene comune, con questa capacità di collaborazione con la capacità di portare a casa risultati. Quindi ringrazio la gestione del Senato fatta in questo modo dai nostri Questori, insieme ovviamente a tutte le altre risorse presenti. Grazie davvero perché questo dà fiducia anche a noi nell'istituzione in cui trascorriamo la gran parte della nostra giornata, e ci permette di sperare che ci possa essere un momento migliore, migliore, in cui talenti e capacità possano trovare le loro occasioni per esprimersi in modo adeguato. Devo dire che i ringraziamenti non possono finire qui. Ho partecipato diverse volte quest'anno agli incontri mensili del sabato promossi dalla

abbiamo la fortuna di invitare per far partecipare persone perché godano dello spessore culturale di quello che è il Senato, affinché capiscano la bellezza della musica in questa Sala; si rendano conto della bellezza della Sala, ma anche delle sue possibilità acustiche. Il che dà l'idea di essere in una istituzione di altissimo profilo culturale. Abbiamo goduto anche - perché no? - di una collaborazione assoluta del personale, di tutti i consiglieri parlamentari e i collaboratori presenti in Aula e qua fuori. dire, se volete un po' sorridendo, che non è mai mancata una mascherina a nessuno di noi perché, prima di entrare in Aula, c'è sempre qualcuno che ci offre una mascherina a tutela nostra e degli altri con la mediazione dell'amabilità e della gentilezza del personale, che è veramente la cifra e lo stile del Senato. Certamente, tutto ciò è molto bello e riempie il cuore di speranza: le più alte istituzioni dello Stato sono in grado di garantire qualità di servizio sotto il profilo umano, scientifico, tecnico e culturale. Cosa ci preoccupa in questo contesto? L'hanno detto anche i colleghi intervenuti prima. Per esempio, ci preoccupa quel personale che, invece, circonda il Senato in condizioni di maggiore fragilità. Penso oggettivamente ai nostri collaboratori parlamentari e non mi riferisco soltanto alla dimensione economica perché sembra che tutto questo si debba tradurre in una contrattualità cui risponde Mi riferisco all'investimento professionale che le persone impegnate in questo ruolo possono avere rispetto alla loro vita.

cento della legislatura. Ne troveremo davanti una parte più ridotta e sappiamo che essa prelude a una sorta di collo di bottiglia, un imbuto perché, se adesso siamo 321, tra un paio di anni i senatori saranno soltanto 200. Cosa ne sarà del personale dei nostri uffici, delle loro competenze acquisite, dello stile di lavoro e del rigore che ha fatto

Che tipo di aspettativa di professionalità in termini di sicurezza, garanzia di competenza, ma anche in termini di tutela di competenze acquisite? Non dimentichiamo che il vero investimento che il Senato fa è nell'acquisire ogni volta nuove competenze. In un certo senso, funziona come una *learning organization*, in cui, di volta in volta, si acquisiscono nuove competenze. Per esempio, tutta la digitalizzazione spinta di questi ultimi mesi ha costituito un arricchimento personale, ma anche istituzionale.

ci aiutano e ci assistono in tanti modi e in tante occasioni. Grazie lo dico mille volte, ma, come collega, lo dico in modo particolare al dottor Marini, che si è preso cura della salute di ognuno di noi sempre e in qualunque manifestazione. *(Applausi)*. Noi vorremmo che davvero, da questo punto di vista, il Senato facesse scuola e fosse un modello di istituzione che garantisce obiettivi, trasmette cultura e, nonostante tutto, è un'oasi di pace in cui si può lavorare bene, serenamente e costruttivamente, cosa che non sempre accade. Signor Presidente, a nome della Lega naturalmente anch'io dichiaro il voto favorevole sia al Rendiconto delle entrate e delle spese per l'anno finanziario 2019, 2019, sia al Progetto di bilancio interno del Senato per l'anno 2020. L'unica osservazione che mi sento di muovere - lo faccio subito - è che forse possiamo migliorare, almeno da un punto di vista, e cercare di arrivare all'approvazione del bilancio

uno dei pochi obiettivi sui quali ancora possiamo lavorare per migliorare. So che il Collegio dei Senatori Questori ha approvato il bilancio, se non sbaglio, a metà anno, verso giugno (mi confermerà o smentirà il questore De Poli nella replica), ma il Consiglio di Presidenza di cui faccio parte l'ha affrontato solo nelle ultime settimane. Cerchiamo, dov'è possibile, di provvedere migliorando da questo punto di vista. È ovvio che la valutazione di un bilancio pubblico che utilizza risorse pubbliche, frutto delle tasse e del lavoro dei cittadini,

Abbiamo apprezzato il fatto che anche quest'anno ci siano dei risparmi, naturalmente per quanto riguarda il rendiconto. È un percorso che è iniziato da lontano, nel 2013; spesso il senatore De Poli cita i quasi 300 milioni di risparmi dal 2013 ad oggi. È ovvio che nella fase iniziale, nel 2013, il margine per risparmiare era elevato, perché si è inciso maggiormente. Man mano che si procede risparmiare su ciò che già si è tagliato diventa sempre più difficile e impegnativo, però auspichiamo che questo percorso non venga interrotto, ma che ogni anno ci sia uno sforzo da parte del Senato migliorare queste prestazioni. *(Applausi)*. Al di là dei risparmi di un'annualità, c'è anche da dire, onestamente, che i senatori in questa legislatura hanno approvato provvedimenti molto significativi in questa direzione, i cui frutti ovviamente non vedremo nell'immediato, ma nei prossimi anni: mi riferisco naturalmente alla revisione del regime dei vitalizi, che è stata

se le sentenze saranno favorevoli, come ci aspettiamo e siamo convinti che lo saranno, vedremo dei risparmi considerevoli per un regime dei vitalizi più equilibrato e più equo. Questo era l'obiettivo, senza penalizzare nessuno. L'altro grande provvedimento che è stato approvato da tutti i senatori, credo da tutti i Gruppi, è la riforma della riduzione del numero dei parlamentari, che in termini assoluti per i bilanci dello Stato rappresentano una piccola cosa, un intervento che sicuramente non risolleverà le sorti del Paese e non inciderà in modo significativo sulla riduzione della spesa pubblica, ma era una questione di principio alla quale tutti noi ci siamo associati in un momento di difficoltà, che purtroppo è diventata ancora maggiore a causa dell'emergenza Covid. Ognuno deve fare la sua parte; noi potevamo incidere in questa direzione e ce ne siamo assunti la responsabilità. Il nostro compito sarà quello di fare in modo che, a fronte di questa riduzione di rappresentanza dei cittadini, quindi parlamentare, il Senato e la Camera sappiano comunque funzionare adeguatamente e in modo anche migliore rispetto al passato. Abbiamo apprezzato i continui investimenti per l'abbattimento delle barriere architettoniche, gli investimenti sul digitale e le infrastrutture informatiche. Da questo punto di vista gli investimenti che sono stati fatti nel passato sono stati evidentemente perché hanno permesso, in questa fase così particolare di necessità di distanziamento, che lo svolgimento dell'attività, soprattutto delle Commissioni, fosse garantito adeguatamente e senza che l'emergenza ponesse problemi o impedimenti. Faccio riferimento anche alla questione, che forse non è stata toccata dai colleghi, dei concorsi per l'assunzione di personale,

dell'istituzione Senato della Repubblica, la sicurezza e la garanzia della salute di tutti noi e soprattutto dei dipendenti che, insieme a noi, non hanno mai lasciato questo Palazzo, neanche durante il *lockdown*. il dottor Marini. Lo hanno fatto già altri, ma anche noi, come Gruppo, sentiamo la necessità di farlo, perché è stata una guida sicura, che ha dato serenità a tutti, con grande professionalità e impegno. Ringraziamo naturalmente anche la struttura e tutti i suoi dipendenti, a partire dagli assistenti parlamentari, e il Segretario generale, Elisabetta Serafin, e tutti i suoi collaboratori, che, al pari di tutti noi, non hanno mai abbandonato quest'Aula e hanno sempre garantito, con la loro professionalità, che i lavori si svolgessero al meglio delle nostre possibilità. *(Applausi)*. Signor Presidente, gentili colleghe e colleghi, vorrei intervenire oggi con una premessa e un auspicio. La premessa riguarda la modalità di approvazione del bilancio interno del Senato ed è fondata su una anomalia, se vogliamo chiamarla così. Ai sensi dell'articolo 165 del Regolamento, il progetto di bilancio e il conto consuntivo delle entrate e delle spese del Senato sono predisposti dai senatori Questori e deliberati dal Consiglio di Presidenza, per poi essere trasmessi al Presidente della 5a Commissione permanente ed infine sottoposti al voto dell'Assemblea: è il voto di oggi. Il progetto cui si riferisce l'articolo 165, che oggi votiamo, è relativo a un bilancio di previsione, come indicato, del resto, nel documento predisposto annualmente dai senatori Questori. Per definizione è un progetto di bilancio preventivo e si riferisce all'esercizio finanziario successivo a quello in cui esso viene redatto e approvato. Tuttavia, la prassi strana, affermatasi negli ultimi anni qui in Senato, va nella direzione diametralmente diametralmente opposta, in quanto il progetto di bilancio preventivo per l'anno 2020 è quella che noi approviamo oggi, a metà dicembre, quando mancano solo due settimane al termine dell'anno. Negli ultimi due anni è successa la stessa cosa: il bilancio preventivo dell'anno contabile in corso è sempre stato approvato alla fine dello stesso e non alla fine del precedente. Concludo questa premessa nella speranza che il bilancio del 2021 lo si possa realizzare entro il primo trimestre o semestre del prossimo anno, così da consentire, a ciascun senatore e all'Assemblea nel suo insieme, di esercitare i poteri di indirizzo in ordine alla programmazione della spesa. Fa piacere che anche il senatore Tosato sia dello stesso parere. Dopo questa premessa, è doveroso intervenire riprendendo il filo di un discorso avviato in quest'Aula lo scorso anno. Da parte dei colleghi senatori Questori, c'è stato un impegno formale ad affrontare il tema della regolamentazione dei nostri collaboratori. Il senatore anziano De Poli affermò in quest'Aula che il Collegio dei Questori avrebbe suggerito in Consiglio di Presidenza di valutare l'opportunità di individuare tipologie contrattuali specifiche e modalità di pagamento per i collaboratori parlamentari, al fine di garantire loro una retribuzione proporzionale e adeguata al lavoro prestato, analogamente all'impegno della Camera dei deputati, nell'intento di trovare una soluzione unica. Aggiungo che lo ha ribadito anche poco fa, in maniera ancora più dettagliata. Quindi, il tema è attenzionato. Capisco che in quest'anno di crisi pandemica, in cui anche l'amministrazione del Senato ha avuto molto da fare, sia stato difficile lavorare su più tavoli, ma credo che la questione debba essere messa all'ordine del giorno del Consiglio di Presidenza quanto prima. Riconoscere la figura del collaboratore parlamentare e disciplinare in modo migliore il rapporto di lavoro con il proprio senatore è un dovere non più rimandabile. Con la storica riforma della riduzione del numero dei parlamentari, da noi fortemente voluta, si si pone ora il tema di normare, insieme alle necessarie modifiche legislative e regolamentari conseguenti alla riforma costituzionale, la funzione che quotidianamente viene svolta dai nostri collaboratori. *Staff* preparati e retribuiti con correttezza e trasparenza saranno ancor più necessari con l'aumento del lavoro per ogni singolo senatore, inevitabile visto che il numero delle Commissioni e degli impegni e rimarrà inalterato. So della presentazione di alcuni disegni di legge certamente da supportare su questo tema, che però può essere risolto semplicemente con un voto in Consiglio di Presidenza. Il Consiglio di Presidenza è il vertice amministrativo del Senato e deve affrontare i problemi e risolvere le questioni rimaste in sospeso da tempo; non può prestarsi a divenire il luogo dove temi scomodi o che non convengono economicamente ad alcuni partiti politici non maturano mai. Colleghi, parliamo quotidianamente dei problemi dei diritti dei lavoratori. Non possiamo permettere che nella casa di tutti gli italiani, dove spesso chi assiste il parlamentare viene sottopagato o retribuito con forme contrattuali inadeguate, questa situazione rimanga irrisolta. Concludo nella speranza - ma sono certo che sarà così - che il Collegio dei Questori lavorerà concretamente su questa tematica, in modo parallelo a quello del lavoro delle Commissioni competenti sui disegni di legge, per arrivare entro la fine della legislatura a una normativa finalmente più trasparente nel rapporto tra parlamentari e collaboratori. Gentili senatori il mio intervento non deve lasciare il tempo che trova. Non sarebbe accettabile assistere ad altri dodici mesi d'inerzia per ritrovarci, nel dicembre 2021, a dover mettere in atto un tira e molla anche solo per la presentazione di un semplice ordine del giorno al bilancio interno. Concludendo, oggi ho il piacere di esprimere la posizione del MoVimento 5 Stelle sul voto del progetto di bilancio interno del Senato, che certamente sarà favorevole. Sono stati svolti buoni lavori in merito all'ottimizzazione delle risorse economiche disponibili. Non posso che compiacermi per l'avvio delle procedure concorsuali per il rinnovo del personale presente negli uffici interni, nuova linfa per l'anima stessa del Senato, personale indispensabile per il corretto funzionamento delle istituzioni. Grazie ancora per il lavoro svolto che, spero, da buono diventi eccellente il prossimo anno.

intervengo oggi perché l'altro giorno ho letto una notizia che mi ha lasciato alquanto perplessa. Vi ricordate quella norma inserita nel decreto rilancio, all'articolo 180, dal titolo "Ristoro ai Comuni per la riduzione del gettito dell'imposta di soggiorno e altre disposizioni Già all'epoca - ed era metà luglio - avevo portato all'attenzione di quest'Aula quello che qualche giornale aveva bollato come "decreto rilancia suocero". L'articolo 180, dietro una rubrica dagli intenti meritevoli, celava ai commi 3 e 4 altre disposizioni, che prevedevano una depenalizzazione del reato di peculato per coloro i quali, proprietari di strutture ricettive quali alberghi e hotel, avessero riscosso la tassa di soggiorno dai clienti e non l'avessero versata al Comune di appartenenza. È ormai noto a tutti che, proprio grazie a questa norma, il signor Paladino, i cui rapporti con l'avvocato Conte sono ben noti, condannato a un anno e due mesi di reclusione proprio perché colpevole di non aver versato la tassa di soggiorno al Comune di Roma nell'arco di tempo compreso tra il 2014 e il 2018 - queste sono parole che ho rilevato dai giornali

Ma tale deputato dovrebbe essere consapevole di aver votato a favore di quell'articolo, dando a suo tempo la fiducia a questo Governo. E se solo oggi si chiede da dove sia arrivata quella norma, gli posso rispondere io, che forse sono stata più attenta di lui ai lavori parlamentari. Arriva da un emendamento "marchetta" - come si dice in gergo - l'emendamento 87.10, presentato dal MoVimento 5 Stelle nella scorsa legge di bilancio, quando il Covid non c'era; un emendamento, già bollato a suo tempo dai giornali con la sanatoria sui reati del suocero di Conte,

All'epoca ero rimasta indignata e lo sono tuttora; se poi anche altri colleghi volessero unirsi all'indignazione, magari potrebbero evitare di regalare la loro fiducia a personaggi che non se la meritano. *(Applausi).*

il mio intervento è teso a rimarcare la gravità di un episodio di violenza urbana verificatosi ad Acerra, un Comune in provincia di Napoli. In questa cittadina la popolazione già vive quotidianamente sulla propria pelle le difficoltà economiche, il degrado sociale e le conseguenze negative di un territorio martoriato da un alto tasso di inquinamento ambientale e da un elevato rischio per la salute, legato sia alla presenza costante e diffusa di roghi tossici della cosiddetta terra dei fuochi, sia alla localizzazione nel suo territorio del termovalorizzatore e dei suoi possibili effetti nocivi. Ebbene, nella notte tra il 12 e il 13 dicembre, ad Acerra sono state date alle fiamme due auto della polizia municipale. Sono ancora in corso le indagini degli inquirenti sulle possibili cause di quanto accaduto. Resta comunque l'assoluta gravità dell'episodio, ove ne fosse confermata la natura dolosa; un gesto di un folle, una vendetta, una ritorsione o, peggio ancora, un atto intimidatorio o, infine, l'idiozia di qualcuno che potrebbe vedere nell'azione di controllo svolta dalla polizia locale, ancor più attenta durante questa pandemia, una limitazione delle proprie libertà, non volendo considerare che queste restrizioni sono giuste e indispensabili per cercare di limitare la diffusione del Covid-19. I cittadini sono indignati e spaventati. L'episodio, qualunque ne sia la causa, rappresenta un segno evidente del degrado e delle grosse difficoltà ambientali e del vivere sociale che accomuna purtroppo tante città del nostro Paese. Sono fiducioso dell'operato e dell'azione della magistratura per una rapida conclusione delle indagini che assicurino alla giustizia il responsabile o i responsabili di questo insano gesto, anche per dare alla comunità un segnale chiaro della presenza e dell'azione costante sul territorio delle istituzioni. Lo Stato c'è.

finestra"), che riguarda il Fondo pensione complementare per i giornalisti italiani, cosiddetto Fondo giornalisti. Gli organi di amministrazione sono caratterizzati da una composizione paritetica, ovverosia da uno stesso numero di rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro; un dialogo tra le parti, fondamentale in questi casi. Da una notizia di stampa apprendiamo che il 23 giugno 2020 il consiglio di amministrazione del Fondo giornalisti ha affidato l'incarico di direttore generale a una persona che ricopriva la carica di consigliere all'epoca della votazione per la sua stessa nomina. Il suo stesso è stato quindi decisivo. Si tratta di una scelta che di fatto mette a repentaglio il dialogo tra le parti - ripeto - fondamentale in questi casi, in un presidio così importante per il *welfare* dei giornalisti italiani. 3, lettera *e)*, dell'Avviso di selezione per l'incarico di direttore generale del Fondo giornalisti, tra le condizioni necessarie per partecipare alla selezione, prevede l'«assenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale». Tale previsione mira a garantire l'indipendenza e la terzietà del soggetto destinato a ricoprire la carica di direttore generale del Fondo. come ragione di incompatibilità, possa esservi anche l'esistenza di una situazione soltanto potenziale di conflitto di interesse.